Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, cari colleghi, siamo quasi in chiusura di una attività legislativa prima della pausa estiva vorrei esprimere fin da subito il mio personale ringraziamento per i lavori della Commissione, unito al convinto voto contrario del Gruppo dei Conservatori Riformisti a questo provvedimento, che non può essere definito con un solo aggettivo, trattandosi di un cattivo decreto-legge e di un pessimo lavoro proposto dal Governo. Pessimo nel merito e nel metodo ma che, comunque, ha visto l'attività della Camera dei deputati e del Senato impegnata nel miglioramento del testo. Secondo noi, però, questo provvedimento costituisce un po' la *summa* dell'idea di Governo, di un Esecutivo la cui attività sembra ormai piegata solo all'opportunismo del momento e alla contingenza dei fatti e degli eventi.

soprattutto molti colleghi, un paio di questioni tutt'altro che di secondo piano e non sono solo di questi giorni: l'assoluto disprezzo per le regole che presidiano l'attività legislativa. Cosa dice l'attuale maggioranza di questo provvedimento? Va tutto bene così? Esattamente come avviene ogni volta l'attività parlamentare è oramai sopraffatta dall'attività legislativa del Governo. quella maggioranza che un tempo faceva grande sfoggio di parole e richiami altisonanti al rispetto delle regole chiedo: non valgono più quelle regole? Cosa dice il Governo

decreto *omnibus* come tanti che continuano a deteriorare l'attività legislativa del Governo e - ahimè - anche del Parlamento. Infatti, il pareggio di bilancio delle Regioni, il dissesto finanziario delle Province, le calamità naturali o quelle indotte dall'uomo, le fondazioni lirico-sinfoniche e le concessioni balneari cosa hanno a che vedere con una visione organica degli enti territoriali ai quali nel titolo questo decreto-legge si rivolgeva? Forse questa eterogeneità è comprensibile alla luce di un altro aspetto inquietante del *modus operandi* di questo Governo, cioè l'assoluta estemporaneità, l'improvvisazione che diventa regola, che diventa legge, ahimè. Il provvedimento in discussione è l'ultimo in ordine di tempo delle ormai innumerevoli prove di quale sia la parola d'ordine dell'azione governativa nel fronteggiare i purtroppo molti e complessi problemi del Paese. La parola d'ordine è una sola: uno *spot* o al massimo un *tweet*. Ecco, quello in esame è un decreto-legge di *tweet*. Questa modalità sta a testimoniare l'inadeguatezza di un Esecutivo che non ha una visione complessiva dei problemi del Paese, quindi non è in grado di creare un tessuto normativo omogeneo e stabile nel tempo attraverso attraverso il quale intervenire per risolvere i problemi. Nel suo armamentario ci sono solo l'emergenza, il rappezzo, il rinvio: mai una risposta puntuale

Cosa rappresentano, infatti, se non un rappezzo, le norme sulle concessioni balneari introdotte nel corso dell'esame alla Camera? Con esse, a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia tenta maldestramente di fare qualcosa per un'annosa vicenda che coinvolge buona parte delle economie territoriali del nostro Paese, ma l'unico vero risultato che ottiene è violare ancora la normativa europea, esponendo probabilmente l'Italia a una nuova procedura d'infrazione che peserà sulle tasche dei nostri concittadini, ovviamente senza risolvere il problema. Invece, alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, margini di trattativa con la Commissione si sono intravisti; tuttavia, per fare questo occorre avere la conoscenza, la competenza e la capacità d'intervenire nel quadro dell'armonizzazione delle normative europee derivate dalla direttiva Bolkestein in modo preciso, capace e funzionale agli interessi della nostra industria balneare, un'industria importantissima,

oggetto invece di continui interventi disorganici e improvvisati che hanno portato a definire una normativa ormai quasi inestricabile. Noi, invece di agevolare la vita delle istituzioni locali, la stiamo complicando ulteriormente. quindi che la meraviglia di fronte alla cosiddetta opinione pubblica che esprime al riguardo un silenzio, che evidentemente va letto come assenso, non deve più stupirci. però dimentico che sono ormai lontani i tempi delle polemiche e dei girotondi; oggi viviamo un'emergenza rappresentata non tanto e non solo dai problemi dei nostri enti territoriali, quanto invece da un Governo che, non potendo affrontare le questioni nel merito, si limita a interventi *spot* e pubblicitari di questo genere, che non aiuteranno alcun ente territoriale ad affrontare la stagione difficilissima che sta davanti a noi, dopo aver indebolito il tessuto delle istituzioni locali. Infatti, si è voluto fare questo proprio nell'ottica di una riforma costituzionale che torna a centralizzare molte competenze, a a far prevalere la vita, le esigenze e le dinamiche dello Stato centrale contro quelle degli enti territoriali, che invece rappresentano una parte fondamentale della storia e della vita pubblica del nostro Paese. Per non solo quello in esame è un decreto-legge che non risolve nulla, ma è una briciola lanciata agli enti territoriali, ai quali verrà tolta non solo competenza, ma anche la natura e il ruolo stesso di presidio più vicino ai cittadini, di realtà istituzionale legata al controllo e alla capacità dei cittadini di poter misurare come, attraverso le loro tasse, vengono erogati i servizi.

è già stato detto tanto sulla questione del metodo nell'affrontare questo provvedimento, ma una cosa che forse sfugge è la ragione per la quale fare questo provvedimento.

definisco allucinante. Della serie: «Aspetta, c'era questo problema, gli metto questa toppa. C'è quest'altro e risolvo in questo modo. Aspetta, ci sono questi scontenti e faccio quest'altra cosa».

ci sono fiducie al Senato e fiducie alla Camera, provvedimenti a iosa, che molte volte vengono approvati e dopo nemmeno due mesi vengono modificati. L'importante è fare: movimentiamo, facciamo fumo, scompigliamo la vita dei cittadini, rendiamo incomprensibile tutto.

Guarda caso, prima erano cose non degne di attenzione: «chi se ne frega dell'alluvione del Veneto; chi se ne frega del terremoto avvenuto in Lombardia e Veneto».

E poi c'è anche il sistema delle Province. Vediamo, all'interno del provvedimento, norme per il dissesto delle amministrazioni provinciali, rideterminazione delle sanzioni, finanziamento delle funzioni fondamentali delle Province. Però, attenzione, chi ha creato il problema alle Province? Chi ha creato questa situazione alle amministrazioni provinciali?

stavamo dicendo cose non vere, cose che vedevamo solo noi; ora però è dimostrato che quanto dicevamo era vero e che il problema era serio. C'è poi la questione dei Comuni:

sanzioni. Chi se ne frega, questo è il concetto. Questo Governo non si è mai preoccupato dei Comuni virtuosi, dei Comuni seri, dei Comuni che amministrano in modo veramente oculato le risorse pubbliche. Chi amministra bene secondo noi va premiato,

Non comprendo, signora Presidente, questo modo di agire. Secondo noi bisogna avere un progetto serio ed organico e non avere, come dicono dalle mie parti, la fregola di farsi vedere. Io sto notando questo e mi dispiace, perché chi ne paga le conseguenze sono i cittadini; il problema ricade su di loro. Stiamo attenti anche alla norma sui minori stranieri non accompagnati, che è un problema serio, serissimo, che molte volte ricade sui Comuni. Però è sottile questo aspetto, perché adesso viene introdotta questa norma, con cui viene dimostrato che i Comuni non riescono a far fronte all'accoglimento di questi minori non accompagnati. E il Governo cosa fa? Dà massima autorità al prefetto (quindi alla lunga mano dello Stato) di disporre le strutture. Ma come, i Comuni dicono che non riescono Chi se ne frega. Il prefetto ha l'autorità di fregarsene di quello che vuole il Comune. Ma chi se ne frega, tanto questo è il sistema utilizzato da questo Governo. Per tutte queste ragioni, noi voteremo contro.

quando ho visto che era stato assegnato ai lavori della nostra Assemblea un decreto che recava nel titolo il sostegno all'azione degli enti locali.

per mancanza di fondi, ma sono diventati l'unico riferimento dei cittadini, il più diretto, il più immediato rispetto alle Regioni e ad uno Stato che si avverte sempre più lontano quando non addirittura

Ciò che emerge, complessivamente, non è soltanto la confusione dell'intervento, la mancanza di organicità e quindi l'incostituzionalità di un decreto-legge che, essendo eccessivamente generico e riguardando settori troppo diversi, non può trovare compatibilità con la nostra Carta costituzionale, ma ancora una volta - e come se ce ne fosse stato il bisogno

questo è il Governo che toglie ai poveri per dare ai ricchi, questo è il Governo che si diverte a farsi bello con le banche, le assicurazioni, le *lobby* più forti che si aggirano non solo nel nostro Paese ma anche nel nostro continente, fregandosene di tutto, annullando del tutto la capacità di rappresentare i bisogni delle nostre categorie e dei nostri cittadini.

dell'accordo istituzionale, che loro avrebbero chiamato di finanza pubblica, tra lo Stato e la Regione siciliana. Sapete cosa è accaduto nella Regione siciliana? nella Regione siciliana? È stato mandato direttamente da Firenze un tale professor Baccei con l'incarico di svolgere il ruolo di assessore regionale alle finanze.

Baccei come Verre a suo tempo - che utilizzano la forza, la determinazione e il potere che viene loro dallo Stato centrale

Hanno fatto un accordo in base al quale, per avere il riconoscimento della stabilità di bilancio per l'anno 2013, si ingabbia del tutto la possibilità di fare manovre negli anni successivi. E si fa anche qui che il tallone dello Stato centrale si fa sentire non solo sull'istituzione Regione siciliana, ma sulla faccia delle siciliane e dei siciliani che oggi vivono un travagliato momento di crisi economica e occupazionale. Il tallone si sostanzia in questo: erano stati avviati diversi contenziosi costituzionali, dal momento che la Regione siciliana doveva ottenere circa 5 miliardi di euro dalle casse dello Stato centrale. Alcuni di questi ricorsi erano già stati vinti.

non si ha il riconoscimento del bilancio 2013 e deve essere dichiarato il *default* della Regione. Tutto questo avviene alla vigilia di una mozione di sfiducia, presentata al

presentato un emendamento che voleva aiutare il Comune di Pozzallo a superare lo stato di *default* e di dissesto. Il Comune di Pozzallo è l'avamposto del nostro Paese nel Mediterraneo, quello che sta compiendo i maggiori sforzi

Qual è questo Governo, che di tale nome possa fregiarsi, che può del tutto disinteressarsi delle problematiche della quotidianità del popolo che, voglio ricordarvi, è sempre sovrano? A questa maggioranza, che sostiene il Governo, che anche oggi si accinge a votare una fiducia

che pagherete un prezzo politico caro. Ai colleghi siciliani voglio dire che non vale fare gli ascari attraversando lo Stretto di Messina e dimenticando l'appartenenza al proprio territorio. Ai colleghi delle altre forze politiche che sostengono il Governo voglio dire che la moralità della politica sta proprio nel fatto di non rinnegare mai ciò per cui si ritiene di aver combattuto. Oggi voi convertire un decreto-legge che è la negazione del programma elettorale che avete proposto al popolo italiano.

Presidente, onorevoli colleghi, la riforma degli enti locali che abbiamo esitato lo scorso anno non poteva che rappresentare un punto di partenza e non di arrivo. Questa è la ragione per la quale sono forse sembrati eccessivi i toni trionfalistici che l'hanno accompagnata, dal momento che prima di esprimere giudizi definitivi è necessario verificare bene l'applicazione pratica. Allo stesso modo, però, non bisogna giudicare negativamente provvedimenti come quello che stiamo esaminando oggi,

materia finanziaria, anche e soprattutto alla luce delle complicazioni riguardanti la nuova architettura degli enti locali e le loro diverse articolazioni. Ecco perché, al di là delle critiche che il provvedimento in esame ha suscitato in quest'Assemblea, mi chiedo come si possano biasimare disposizioni che, di fatto, tendono a far respirare i Comuni, incidendo sul Fondo di solidarietà comunale per quegli enti che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI e per i quali vengono accantonati 80 milioni di euro. alle disposizioni previste per i Comuni emiliani colpiti dal sisma del 2012, o - ancora - alla previsione del differimento di alcuni termini a favore di Comuni che rischiano il dissesto per sostenere spese per condanne di risarcimento relative ad eventi calamitosi e, ancora, le norme per facilitare il risanamento degli enti che abbiano già dichiarato il dissesto. Allo stesso modo, mi chiedo come non apprezzare le disposizioni con riguardo ai vincoli di bilancio, che prevedono l'attenuazione delle sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015. È altresì degna di nota l'istituzione del Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni, con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il triennio 2016-2018. Si è parlato di provvedimento *omnibus* e *spot*, ma non dimentichiamo che tante norme sono il frutto dell'accoglimento di talune istanze delle Regioni e dei sindaci. Cito, per esempio, l'articolo 10, con il quale vengono recepite le numerose proposte normative presentate dalle Regioni concernenti la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome. Qualcuno ha invocato la necessità di leggi più organiche. Sono d'accordo, quando queste si possono fare. Non dimentichiamo che, specie negli ultimi anni, in fatto di misure finanziarie per gli enti locali bisogna purtroppo fare i conti con delle contingenze emergenziali. Guai se ce lo scordassimo, perché sottovaluteremmo il fatto, ad esempio, che i Comuni sono soggetti alle loro scadenze e che devono osservare le loro regole, per esempio in materia di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione di opere in compartecipazione a valere su fondi comunitari. Potrei dilungarmi ancora su questo argomento. questo per segnalare che è giusto che, quando se ne ravvisi la necessità, il Governo faccia fronte alle esigenze dei territori con provvedimenti che a taluni possono sembrare deprecabili o utili solo per operazioni mediatiche. Personalmente, non ne sono convinto. La pianificazione e la programmazione devono essere la bussola per ogni amministratore, ma è altrettanto indice di buon governo e buona amministrazione avere la giusta dose di flessibilità per fronteggiare situazioni sempre nuove o che richiedono risposte nuove. Certo, convertire decreti-legge a pochi giorni dalla sospensione estiva non è cosa auspicabile, dal momento che, motivato dalla necessità di scongiurare ulteriori passaggi navetta tra Camera dei deputati e Senato, il Governo ha ritenuto di dover ricorrere al meccanismo della fiducia per non paralizzare il percorso. Questo reca con sé, inevitabilmente, un *vulnus* per le facoltà emendative dei parlamentari, che sono impossibilitati a far inserire correttivi ed emendamenti migliorativi del testo. Ma va da sé che quando non c'è altra alternativa, se non il rischio di spiaggiamento del provvedimento per l'incombere delle ferie estive, bisogna aderire senz'altro alla teoria del cosiddetto male minore. Poiché sono persuaso della bontà di alcune disposizioni contenute del provvedimento che alcune di esse sono ampiamente attese dai Comuni, Province e Regioni, sono convinto che talune avranno certamente un impatto positivo nei territori. Ritengo che, nel caso specifico,

il testo sul quale il Governo ha posto la fiducia è certamente corposo e contiene un insieme di misure destinate agli enti territoriali che apparentemente possono sembrare disorganiche, ma che vanno invece lette in un contesto più ampio, ossia insieme a quei provvedimenti sui quali abbiamo lavorato in questi ultimi tempi quali, solo per citarne alcuni, quello sull'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e la legge di stabilità per il 2016. Nel provvedimento Nel provvedimento è stato individuato, a nostro avviso, un punto di equilibrio ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, e dunque in ordine al Patto di stabilità interno, al pareggio di bilancio, al Fondo di solidarietà e definizione del contributo degli enti locali. La questione di fiducia posta dal Governo non è stata quindi motivata esclusivamente da ragioni di urgenza, seppure esistenti, ma dall'esigenza di impedire un complessivo stravolgimento del provvedimento, così come approvato in prima lettura alla Camera. Sotto il profilo strutturale, quelle del provvedimento costituiscono misure urgenti ai fini del risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità e la previsione di poter ricorrere ad una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali ove siano presenti squilibri di bilancio così rilevanti da poter provocare un dissesto finanziario. Si concorre in tal modo, anche con la riforma del bilancio, ad un percorso virtuoso degli enti locali, sulla base di indirizzi che certamente devono essere flessibili in ordine alla diversità delle situazioni esistenti. Ma nel contempo si introducono parametri uniformi, di sistema, sul piano nazionale e si determina, sempre entro un quadro di compatibilità, di restituire agli enti locali, in primo luogo ai Comuni medi e piccoli, alcune capacità gestionali, ad esempio con margini di manovra, in parte anche al di fuori dei tetti di spesa, per quel che riguarda la assunzione del personale, con particolare attenzione al *welfare* ed al lavoro flessibile. In merito all'attenuazione delle sanzioni previste a carico dei Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità riteniamo che i casi andrebbero valutati con attenzione al fine di evitare che vengano premiate amministrazioni che palesemente hanno disatteso più volte i vincoli imposti da una corretta gestione. Nel corso dell'*iter* in prima lettura il provvedimento è stato integrato e migliorato, anche se alcune questioni rimangono ancora aperte. Riconosciamo, ad esempio, che è stata prevista anche una parziale compensazione della perdita di gettito delle accise dal 2011 al al 2014, nei confronti ad esempio della Regione Val D'Aosta. Mentre, come autonomie speciali, in particolar modo come Province autonome di Trento e di Bolzano, abbiamo posto l'esigenza di ribadire, in fase di attuazione, ciò che è stato definito sulla base delle intese raggiunte fra Governo, Regioni e Province autonome, in relazione al concorso al riequilibrio finanziario e per ciò che attiene agli obiettivi posti dalla legge costituzionale sul pareggio di bilancio. Il confronto con il Governo ha avuto quale esito l'individuazione della legge di bilancio triennale 2017-2019 quale sede, come affermato dal ministro Padoan, «nella quale il Governo si impegna ad affrontare anche le soluzioni proposte dalle Province autonome di Trento e Bolzano per l'utilizzo - secondo le procedure e con i limiti derivanti dagli obiettivi generali di finanza pubblica - degli avanzi presenti nei loro bilanci». Il Governo ha condiviso l'impostazione e le ragioni di merito che abbiamo posto sotto un profilo sostanziale, sulla base della considerazione che «con la riforma della legge n. 243 del 2012, già approvata dal Senato ed attualmente in discussione alla Camera, si è stabilito che dal 2020 il Fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa entri nel saldo delle autonomie locali». La medesima legge, come ha sempre precisato il Governo, prevede che la prossima legge di bilancio per il triennio 2017-2019, che sarà presentata alle Camere entro il 20 ottobre, regoli la transizione nei tre anni che ci separano dal 2020, stabilendo qualità e quantità della progressiva introduzione nel saldo del Fondo, in modo che risulti compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica. Voglio sottolineare proprio questo aspetto specifico, perché si tratta di un elemento che riteniamo essenziale, soprattutto per la ripartenza degli investimenti nei nostri territori. Confidiamo pertanto nelle parole del Ministro e nella rapida soluzione della questione sollevata dalle due Province autonome. Per tutte queste ragioni, ma anche per l'importanza di molte misure previste nel testo in esame, il Gruppo per le Autonomie - PSI-MAIE esprimerà il voto a favore della fiducia.

suo contenuto, abbastanza confuso, come abbiamo avuto modo di dire nel corso

alle misure straordinarie di accoglienza. Si parla ancora di misure straordinarie di accoglienza, di fronte ad un fenomeno che non è straordinario, ma ha una dimensione ormai ordinaria ed è destinato, in ragione delle vicende che riguardano le zone colpite da eventi bellici nella sponda Sud del Mediterraneo e nel Medio Oriente, a crescere ulteriormente e ad essere ancora più costante nel tempo. tempo. Non si può pensare che, attraverso un provvedimento di questa natura, si intervenga a regolare le modalità di accoglienza di persone particolarmente fragili, vittime di pesanti violenze, violenze, psicologiche e materiali. Si deve fare di più e si deve fare meglio: si deve approvare cioè un provvedimento

consentire a questo Occidente così civilizzato da avere la pretesa di esportare i propri costumi politici di governo della società, e a questa Europa antica e così colta, di fare il proprio dovere

si pone il voto di fiducia dopo l'esame alla Camera, spesso mortificando quest'Aula e quest'Assemblea, le sue Commissioni e gli stessi senatori, parlamentari a pieno titolo costituenti quest'Assemblea. Lo si fa ammazzando la discussione all'inizio, cioè non passando neppure attraverso quell'esame, che spesso ha animato la discussione in Parlamento, sugli emendamenti per capire se sia possibile, in ogni caso, migliorare il provvedimento, almeno in parte, e giungere al voto di fiducia solo in presenza di una contrapposizione di natura politica tale da cadere in ostruzionismi inaccettabili. Invece qui la straordinarietà delle procedure viene ripetuta in modo ordinario, manifestando in modo ormai inequivocabile una crisi profondissima del nostro sistema politico parlamentare, una crisi di comportamenti istituzionali inaccettabili, anche attraverso l'esame, che è d'obbligo e che deve essere fatto dal Parlamento e anche da questa Camera, sulla costituzionalità delle procedure e dei provvedimenti, sul rispetto dei capisaldi di finanza pubblica richiamati nella Costituzione, in particolare all'articolo 81. Qui si viola più o meno tutto. Si viola sul piano delle procedure, si viola sul piano delle relazioni politico istituzionali tra maggioranza e minoranze, si viola anche sotto il profilo finanziario, quello che avrebbe dovuto essere il terreno sul quale maggiore controllo viene effettuato. E lo si fa - badate bene all'indomani dell'approvazione delle nuove norme di bilancio e di contabilità pubblica. E questo lo si fa lo dico perché bisogna esserne assolutamente consapevoli - non perché qui ci sono un Parlamento e minoranze che si pongono in netto e sistematico contrasto con le proposte della maggioranza e del Governo.

Lo si fa all'indomani di una approvazione larga, comunque di astensione politicamente significativa, anche su altri provvedimenti. Lo si fa proprio nell'idea che il Parlamento debba subire questo tipo di violenza e la debba subire passivamente, senza poter contribuire con le intelligenze e le capacità che ha alla elaborazione di provvedimenti più adatti più adatti alle esigenze e alla crisi che questo Paese attraversa. Ecco perché, signor Presidente, noi voteremo contro il voto di fiducia al Governo su questo provvedimento. Onorevoli colleghi, sono le ore sono le ore 10,25. Ricorre oggi il trentaseiesimo anniversario della strage di Bologna, uno dei più drammatici attentati terroristici perpetrati in Italia dal dopoguerra. L'ordigno esplose proprio a quest'ora, alle 10,25 del mattino, nella sala d'aspetto della stazione centrale. Si contarono 85 morti e oltre 200 feriti. Le immagini di ampia e violenta devastazione sono impresse nella nostra memoria per sempre. Ancora una volta, dopo la strage del treno Italicus del 4 agosto 1974, le istituzioni e i cittadini si trovarono uniti nello sforzo comune di preservare l'ordine costituzionale e la legalità, mentre vivevano momenti tra i più difficili della storia della Repubblica. Anche grazie al tenace e decisivo contributo dell'associazione dei famigliari delle vittime, ebbe inizio, nel 1987, un lungo percorso giudiziario per accertare la verità sulla strage. La prima condanna definitiva per gli esecutori materiali e gli ufficiali accusati di depistaggio delle indagini si ebbe con la sentenza n. 21 della Corte di cassazione a sezioni unite del 23 novembre 1995.

una risposta di verità e di giustizia sugli intrecci opachi e torbidi che hanno causato morti innocenti e ostacolato la ricostruzione definitiva della strage. Come ha sottolineato il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage, Paolo Bolognesi, è sicuramente importante che proprio oggi entri in vigore la legge n. 133 del 2016, che introduce nel codice penale il reato di depistaggio, nonché una specifica circostanza aggravante per il caso in cui il depistaggio sia commesso in relazione a procedimenti penali relativi ai delitti contro la personalità dello Stato, delitti di strage e di terrorismo. Credo che quest'intervento legislativo, del quale la stessa associazione si è fatta tenace promotrice, possa essere considerato il risultato della piena collaborazione tra il Parlamento e tutti i cittadini che, come nel caso dei famigliari delle vittime e dei testimoni che hanno aiutato la ricostruzione della verità, hanno costantemente offerto alle istituzioni, con coraggio e senso dello Stato, il proprio contributo per la ricerca della verità. Desidero rinnovare la vicinanza del Senato e mia personale a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame risulta essere molto complesso. Esso è il frutto di una lunga attività emendativa svolta alla Camera dei deputati, che sottolinea la necessità di come vada presa in seria considerazione e risolta la situazione degli enti locali. Credo che in questa legislatura su tale situazione siamo stati attenti e abbiamo legiferato diverse volte. La direzione di marcia dell'azione del Governo e del Parlamento era già stata ben delineata con la legge di stabilità 2016, la quale ha segnato la fine dell'epoca dei tagli e il superamento del vecchio Patto di stabilità interno con il pareggio di bilancio. Con le modifiche alla legge n. 243 del 2012, già approvate dal Senato la scorsa settimana, superiamo oltretutto un quadro di regole inapplicabili sul pareggio di bilancio degli enti locali che sarebbero entrate in vigore dal 2017, dando invece continuità alle regole della legge di stabilità 2016 e creando le condizioni per mettere mano al testo unico degli enti locali e in quella sede affrontare le questioni ordinamentali ancora aperte per andare nella direzione dell'autonomia, della responsabilità e della semplificazione. Con questo decreto-legge aiutiamo gli enti locali, miglioriamo la loro situazione contingente. Il provvedimento si pone come un intervento manutentivo dell'ordinamento su alcune questioni che sono in divenire. Diversi sono i punti salienti. C'è una definizione precisa della transizione verso l'abolizione completa delle Province: abbiamo la necessità di garantire, in attesa della riforma costituzionale, alcune funzioni delle Province, che si stanno indebolendo dal punto di vista amministrativo. Su questo provvedimento - ricordiamo - ci sono 100 milioni di euro del Fondo ANAS per la manutenzione straordinaria delle strade, è una funzione importante delle Province. Sono fondi in conto capitale: è un particolare drammatico, se voi andate a vedere l'evoluzione della dinamica della spesa, la spesa in conto capitale di questi anni degli enti locali e della pubblica amministrazione in generale. Per le Province si sono abolite le sanzioni per il Patto di stabilità 2015. La stessa cosa è stata fatta per le Città metropolitane, che sono realtà istituzionali nascenti e su cui c'era stato anche un forte impegno con l'ANCI: anche qui, sul sistema delle sanzioni, c'è l'esclusione delle Città metropolitane per lo sforamento del Patto di stabilità relativo alle competenze 2015. Per quanto riguarda le realtà comunali, anch'esse in una fase di transizione legislativa, voglio ricordare che i Comuni hanno subito la stretta più forte in questi otto anni di politiche di rigore di finanza pubblica; non a caso, sono stati sottoposti ad un Patto di stabilità che spesso è stato considerato irragionevole. Superato il Patto di stabilità previsto per il 2015, siamo nel 2016 in fase di pareggio di bilancio: è quindi anche questa una transizione; per gli enti locali abbiamo attenuato di molto le sanzioni, ad esempio, portandole al 30 per cento dello sforamento ed escludendo dal sistema delle sanzioni le spese che competevano all'edilizia scolastica, che tutti abbiamo considerato una priorità. Per i Comuni è prevista anche una deroga sulle assunzioni per il personale degli asili nido e delle scuole per l'infanzia, ci sono dei contributi per la ritrattazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, sul pagamento delle penali e delle more. Per tutti gli enti territoriali vi è un miglioramento delle norme sul dissesto e pre-dissesto. In materia di personale, per il *turnover* si passa dal 25 al 75 per cento per i Comuni sotto i 10.000 abitanti abitanti virtuosi nel rapporto dipendenti-popolazione e si sblocca la mobilità nelle Regioni dove è stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle Province. Sono stati apportati interventi manutentivi anche su quelle norme che avevano messo in piedi altri Governi, sulle situazioni legate al sisma dell'Emilia e dell'Aquila: ci sono ulteriori 16 milioni di euro per il Comune dell'Aquila, e ulteriori risorse per i Comuni fuori cratere, che pure hanno subito danni e che forse, a volte, vengono messi un po' in ombra rispetto alla centralità aquilana. Comunque, anche qui norme che hanno risposto ad esigenze di quei territori che si erano fatti sentire. Così come è stato inserito nell'ordinamento l'accordo importante, storico, con la Regione Sicilia, che porta alla Sicilia un vantaggio nel meccanismo tra riscosso ed accertato della compartecipazione IRPEF. Oggi la Regione Sicilia può vantare il contributo di 1,4 miliardi di euro Il decreto-legge definisce ulteriormente il *restyling* delle fondazioni lirico-sinfoniche, alcune delle quali rappresentavano un'emergenza, in quanto incagliate nei cosiddetti percorsi di risanamento; ora garantiamo una maggiore flessibilità. Voglio dire, Presidente, che sulle fondazioni lirico-sinfoniche forse la maggioranza e il Parlamento devono fare un'ulteriore riflessione, perché il sistema delle fondazioni non è sostenibile nell'assetto attuale, quindi è inutile che continuiamo a fare interventi tampone. Durante l'esame parlamentare, sono stati introdotti argomenti nuovi, che credo siano patrimonio di tutto il Parlamento: l'ulteriore possibilità di rateizzazione del debito verso Equitalia, che va ad aiutare imprese e famiglie che si sono trovate in difficoltà e che non riescono a sostenere precedenti piani di rateizzazione; si è garantita, in tal modo, un'ulteriore *chance* a quei contribuenti che hanno difficoltà. Così come la soppressione delle tasse aeroportuali è importante per salvare molti aeroporti e per lasciare linee *low costo* che altrimenti andrebbero via. Inoltre, l'assunzione di ulteriori 400 vigili del fuoco è un ottimo segnale a tutela dei nostri patrimoni e per la sicurezza dei nostri cittadini. Per la prima volta viene istituito un fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. Vi sono norme che aiutano ad affrontare l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che aiutano i Comuni colpiti dal sisma di Emilia, Lombardia e Veneto per il pagamento di tasse e contributi relativi a quel terremoto, per le vittime dell'alluvione di Sarno e per le famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato. Finalmente siamo riusciti a stanziare gli indennizzi in favore delle persone affette da sindrome da talidomide, di cui da tempo stiamo discutendo e che ha visto l'impegno di tutti i Gruppi parlamentari. Infine, in merito alla disciplina per gli stabilimenti balneari, abbiamo approvato una norma ponte che ci consente di andare a una legge quadro, su cui il Governo si è impegnato in Parlamento direttamente, che possa consentire di avere una proroga, un periodo transitorio, e andare a una evidenza pubblica che però sia connotata dal recepimento della qualità degli investimenti, del valore degli investimenti fatti dagli operatori balneari e anche della loro professionalità. Insomma, nel provvedimento che oggi approviamo ci sono novità positive per gli enti territoriali, per le attività e le imprese di alcuni comparti produttivi, per il rafforzamento di alcuni servizi importanti della pubblica amministrazione, ma soprattutto per i cittadini. Per tutti questi motivi, signor Presidente, il mio Gruppo, Area Popolare, voterà a favore di questo provvedimento e

senza un confronto appropriato e serio. Ormai sono note a tutti le disposizioni in esso contenute: dal Patto di stabilità interno al Fondo di solidarietà comunale, alle misure per i territori soggetti a calamità naturali e agli interventi per gli enti in crisi finanziaria, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, nonché misure in materia sanitaria, ambientale e agricola. Tra le novità troviamo anche la riapertura della rateazione dei debiti fiscali: per i contribuenti che alla data del 1° luglio 2016 sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari è prevista la possibilità di essere riammessi ad una nuova dilazione, presentando apposita richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto-legge. Questo significa che la chiacchierata soppressione dell'ente di riscossione da parte del Governo non è reale, ma è un'ulteriore proroga dell'abolizione di Equitalia: l'ennesimo rinvio, una storia che dura da quattro anni. con questo provvedimento viene stabilito che gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio consolidato entro i termini di legge non potranno assumere personale, né stabilizzare i lavoratori che già collaborano con loro. Ma quali sono i motivi che inducono gli enti ad approvare tardivamente i menzionati documenti? Negli ultimi anni è diventata una vera e propria tendenza quella della posticipazione dell'adozione della delibera di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ordinariamente prevista entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente. Si tratta di una tendenza che si è ormai consolidata, laddove inizialmente i differimenti erano circoscritti al primo trimestre dell'esercizio finanziario; di recente, invece, essi hanno superato la prima metà dell'esercizio, così riducendo la fase della programmazione sempre più ad un mero adempimento formale. Se i motivi, quindi, risiedono nel fatto che manca la delibera, a questo punto vuol dire che manca la volontà politica; il che è preoccupante, perché così facendo si continua a tralasciare la fase della programmazione, essenziale per decidere su cosa investire, come investire e con quali soldi investire. L'assenza della programmazione vanifica il ruolo stesso del bilancio preventivo ed espone gli enti locali al rischio di esiti gestionali negativi. del patologico prolungamento dell'esercizio provvisorio sull'attività gestionale di ciascun ente, dobbiamo avere il coraggio di dire che essi sono il frutto del Patto di stabilità e del pareggio di bilancio. Sono proprio questi ad avere causato il disastro degli enti locali, in particolare dei Comuni. Nonostante si dica che il Patto di stabilità è stato superato, resta il fatto che questo, unitamente all'equilibrio di bilancio, sta sempre più comprimendo la possibilità per i Comuni di erogare servizi ai cittadini. L'obbligo di pareggio nel bilancio di previsione garantisce ai cittadini che l'ente comunale non spenda più di quanto ha a sua disposizione e allo stesso modo obbliga il Comune a programmare interamente come intenda disporre delle risorse a favore dei cittadini. Ma quale può essere oggi la capacità di spesa di un Comune se si vede sempre più stringere la cinghia? Non è normale che un cittadino non possa più godere del servizio idrico o del trasporto pubblico in maniera efficiente solo perché il Comune dove risiede ha un buco di bilancio! Buco, tra l'altro, non sempre dovuto a cattivi amministratori. Oggi i Comuni sono quelli che più di tutti stanno pagando il consolidamento dei conti dei Governi. I sindaci, ogni giorno, devono lottare contro il grave mostro costituito dall'elevato grado di incertezza sulle entrate proprie di natura tributaria, incertezza dovuta alla difficoltà per i cittadini di pagare la bolletta della spazzatura o l'IMU. Quello che sappiamo è, però, che questo Governo strozza alcuni Comuni e ne salva altri, consentendo di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario. E, infatti, il decreto-legge, all'articolo 15, consente ai Comuni che sono sull'orlo del dissesto di presentare un piano di riequilibrio di bilancio, ma soprattutto di rimodularlo o riformularlo. In effetti, in un decreto-legge onnicomprensivo, che include di tutto, non potevamo che aspettarci qualche sorpresa. Ad esempio la norma su Catania. La scure del fallimento dell'azienda Comune, sembra allontanarsi definitivamente visto che il decreto-legge prevede la proroga dal 30 giugno dal 30 giugno al 30 settembre del termine per presentare, appunto, il piano di rientro, nonché la possibilità di operare in regime di deroga rispetto al testo unico degli enti locali, laddove si parla di approvazione del disavanzo e dei debiti fuori bilancio. Deroga per favorire qualcuno piuttosto che un altro. Solo che ogni volta che deroghi ad una regola, praticamente la cancelli. Questo decreto-legge continua a non risolvere i tanti problemi aperti dalle scelte del Governo in tema di tagli agli enti locali, in particolare alle Province e alle Città metropolitane, e non salvaguarda certo la comunità dei cittadini. E qui mi tornano in mente le parole di Leonardo Sciascia: «La sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei cittadini». Oggi l'opposizione subirà l'ennesima questione di fiducia, ma la fiducia o è piena o non esiste! Per noi non esiste. Anticipo quindi il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle. Signor Presidente, ci troviamo innanzi alla cinquantatreesima fiducia posta da questo Governo al Parlamento nei suoi due rami

e, conseguentemente, neanche una sua strategia complessiva di dialogo con il Paese. Il provvedimento doveva essere censurato *ab origine* per tutti i suoi difetti costituzionali dalla pluralità degli argomenti, alla palese violazione di alcune norme costituzionali. In sede di discussione sulle questioni pregiudiziali ho ampiamente illustrato i motivi dell'incostituzionalità dell'articolo 11, che riguarda l'intesa tra Governo

proposti al Parlamento sotto forma di regole generali che, in realtà, riguardano specifiche esigenze. Ringrazio la relatrice, la senatrice Zanoni, che puntualmente svolge il compito di portare a sistema le norme sugli enti locali. Ciò è però vanificato sia dalla proposta iniziale del Governo, sia dagli inserimenti effettuati alla Camera, sia infine dal fatto che i suoi buoni propositi e la nostra assoluta disponibilità a intervenire assieme sull'argomento, alla fine, si substanziano in ordini del giorno, perché il Senato non ha il diritto, la facoltà, la possibilità di poter apportare modifiche a quanto stabilito prima dal Governo e poi dalla Camera in sede di prima lettura.

non abbiamo più la possibilità di intervenire sui testi normativi, nonostante la buona volontà anche di parte della maggioranza e ci si deve limitare all'elaborazione di alcuni ordini del giorno, che lasciano il tempo che trovano e che, comunque, manifestano una grande insofferenza da parte di tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, sull'impossibilità di costruire un percorso logico, razionale e coeso per quanto riguarda la politica degli enti locali del nostro Paese. Ancora una volta non viene posto alcun argine al differimento delle date di approvazione ormai, la prassi è che i nostri Comuni approvino i loro bilanci di previsione, bene che vada, nell'ultimo mese di vigenza dell'anno di riferimento. approvano il bilancio di previsione a gennaio con riferimento all'anno precedente. Non si riesce ad ottenere dal Governo una discussione organica su queste materie e, quindi, non si riesce neanche a farlo in Parlamento. La necessità del Governo di andare al voto di fiducia dipende quindi dal fatto che

proposito - ben 120 milioni di euro a otto Fondazioni lirico sinfoniche d'Italia indebitate per cattiva gestione dei loro consigli d'amministrazione, diretta emanazione dei Comuni

assolutamente inaccettabile non tanto di singole norme, ma dell'intero contesto che, come dicevo, non porta all'elaborazione di una progettualità definitiva per la gestione dei Comuni e mette in difficoltà gli amministratori e, ancor di più, i cittadini.

e non per tributo e, quindi, se il tributo rimane inalterato, crescono enormemente le tariffe. Inoltre, molto spesso la crescita delle tariffe non corrisponde a un'esigenza del servizio, ma finisce per alimentare un bilancio, che diviene deficitario appunto perché i tributi locali non sono più sufficienti a sopperire ai continui tagli

viene chiesto di fare salti mortali per far quadrare i bilanci e vengono imposti limiti nell'utilizzazione dei loro fondi con forti sanzioni, che poi l'anno successivo vengono tolte e modificate, a seconda di chi

per i nostri enti locali, cosa che questo Governo dimostra di non essere in grado di fare, continuamente e costantemente, e tale decreto è una riprova di questa assoluta incapacità. È per questo e per tanti altri motivi

*(PD)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, senatori e senatrici, il decreto-legge in esame è stato ampiamente modificato nel dibattito alla Camera durante l'*iter* di conversione; al Senato, nonostante i tempi stretti, abbiamo fatto una discussione molto approfondita in Commissione bilancio, di cui troviamo una traccia importante nell'ordine del giorno approvato. Molte misure di questo decreto-legge riguardano gli enti locali, per sostenerli nelle loro problematiche attuali, che non sono semplici. In particolare, vi si trovano disposizioni in materia di Fondo di solidarietà comunale, si stanziano risorse per i Comuni e le zone colpite da calamità naturali

Per le Province, in particolare, affinché possano far quadrare i bilanci, vengono stanziati 148 milioni nel 2016, di cui 100 finalizzati alla loro missione fondamentale, insieme alle scuole, ossia alla manutenzione straordinaria delle strade, e i restanti 48 milioni destinati ad altre funzioni. Sono poi introdotte delle norme finalizzate a promuovere interventi di risanamento per gli enti locali in dissesto finanziario mediante la concessione di anticipazioni di liquidità da restituire in base a piani di ammortamento. A tal fine viene stanziato un contributo triennale di 150 milioni per i Comuni, le Province e le Città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto dal 2011 al 2015, e un contributo di pari importo per il biennio che va dal 2019 al 2020. Viene allentato il blocco del *turnover* nei Comuni fino a 10.000 abitanti e, quanto al personale insegnante ed educativo di scuole dell'infanzia ed asili nido, è stata varata una disposizione che autorizza i Comuni a procedere a un piano straordinario di assunzioni, che vale anche per i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2015. Si istituisce per la prima volta un Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. con l'articolo 9-*ter*, su 136 milioni nel triennio 2016-2018. Come si vede, contrariamente a quanto ascoltato nel dibattito, non si tratta di interventi

e si definiscono le modalità del loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Per le Regioni sono state affrontate anche le questioni della tempestività dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario della spesa farmaceutica, affinché le medesime possano effettivamente recuperare le risorse iscritte nei bilanci (e quindi possano redigere i bilanci). Si dà poi attuazione attuazione all'accordo con la Regione Valle d'Aosta e si mantengono gli impegni con la Regione Siciliana con un patto che prevede impegni reciproci tesi a dare stabilità alle risorse per questa Regione. Se vogliamo individuare una chiave di lettura di questo provvedimento, essa va

cerealitico e lattiero-caseario, settori in cui la crisi ha reso urgenti gli interventi. Voglio concludere però con una riflessione più generale sul provvedimento Si tratta di un provvedimento non casuale, che trova una sua precisa collocazione nel processo di riforma in atto del sistema degli enti territoriali. Voglio solo ricordare in questa sede due importanti provvedimenti, conclusi negli ultimi mesi: il superamento del Patto di stabilità per gli enti locali con la legge di stabilità dello scorso anno e, proprio qualche settimana fa, il disegno di legge di modifica

è la soluzione delle problematiche che emergono nell'attuale situazione, in cui si deve trovare, in particolare per gli enti locali, le Province e le Città metropolitane, un difficile equilibrio tra le esigenze della riforma, che vengono ben messe in evidenza dai provvedimenti attuati, e i severi vincoli di finanza pubblica. Non si tratta quindi di provvedimenti confusi, - come abbiamo sentito dire - o alla ricerca di consenso, quanto di esercizio faticoso ma necessario di responsabilità di governo, per far avanzare un processo di riforme reali e proprio per questo bisognoso di interventi progressivi, anche per sostenere momenti di difficoltà e problematiche e per correggere eventuali errori. Una parte importante di queste problematiche è stata affrontata nel provvedimento altri problemi rimangono aperti, soprattutto per dare certezza e sostenibilità ai bilanci dei nostri enti territoriali e in particolare alle Città metropolitane e alle Province, oltre che ai Comuni e alle Regioni. Su questi temi continueremo ad operare, perché resti molto alta l'attenzione del Governo. Come ho ricordato in precedenza, la Commissione bilancio ha approvato all'unanimità, quindi con il voto di tutti i Gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, un ordine del giorno molto puntuale, che mette questi temi, relativi ai provvedimenti ulteriori da realizzare in questo processo di riforma, al centro dell'iniziativa del Governo e del Parlamento, a partire dalla prossima legge di bilancio. Per questi motivi, quindi, per l'importanza del decreto-legge in esame, per l'importanza di sostenere gli enti territoriali, per l'importanza di dare corso e continuità

Onorevoli colleghi, in relazione all'andamento dei lavori, avverto che la seduta dell'Assemblea, a conclusione della votazione sulla fiducia, sarà sospesa fino alle ore al fine di consentire alle Commissioni di convocarsi e completare l'esame dei provvedimenti in calendario, anche in relazione alla richiesta di alcuni Gruppi di tenere le proprie riunioni.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2495, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, nel testo approvato

Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in aula pone nuovamente al centro del dibattito politico il tema del cibo, in linea con il contenuto ereditato da Expo 2015, "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita", come il simbolo del paradosso che meglio rappresenta le contraddizioni del nostro tempo. L'eccesso e la scarsità, il troppo e il niente, lo spreco e il risparmio, l'egoismo e il dono, la fame e l'inappetenza, la povertà e la ricchezza. Sono i paradossi di un modello economico ed etico che ha disegnato gli squilibri enormi di un mondo ove in alcune parti si acquistano beni e, in particolare, si acquista cibo, ma non sempre lo si consuma più spesso lo si trasforma in rifiuto producendo danni all'ambiente e costi economici e sociali per le comunità e, in altre parti, non si consuma perché il cibo non c'è e spesso non si riesce a produrre nulla e l'impossibilità di alimentarsi domina i pensieri e le azioni dell'intera esistenza. Un mondo in cui 800 milioni di persone soffrono per la fame e altrettanti di eccesso di nutrizione. Nella storia recente della nostra civiltà, lo sviluppo economico ha messo la fame al bando dalle nostre città, dalle nostre campagne, dalle nostre vite, vite, come i vaccini hanno fatto sparire molte malattie. La fame però non è sparita dalle zone più degradate, più marginali, più povere l'abbiamo semplicemente allontanata. I modelli di produzione e di consumo hanno progressivamente modificato finalità e funzioni del cibo come bene primario. La sua utilità non è più stata la variabile principale di quantificazione del valore ma sono entrate in campo altre determinanti, come il prezzo. Ciò fino a quando la crisi non ci è piombata addosso e ha riattivato le categorie sociali della povertà e dalla mancanza di cibo, di nuovo, chiaramente visibili anche dove non c'erano più da decenni. Questo brusco e per di più inaspettato cambiamento sta modificando le scelte di acquisto e le modalità di consumo per molti, aprendo riflessioni e interessi anche sulle abitudini e sui comportamenti portando in superficie quei paradossi con cui il nostro tempo e noi tutti cominciamo a fare i conti. E di numeri se ne stanno raccogliendo tanti. L'Osservatorio Waste Watcher, ad esempio, ha stimato il fenomeno dello spreco alimentare nel nostro Paese e i risultati sono sconcertanti: più di 5 milioni di tonnellate di prodotti alimentari finiscono, ogni anno, nella spazzatura. Si parla di una cifra intorno agli 8 miliardi di euro, mezzo punto di PIL. Le nostre 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari comprendono tutto quel cibo che viene realizzato, trasformato, distribuito e preparato per la somministrazione ma che per diverse ragioni non viene venduto o consumato. Esse si formano per il 57 per cento presso operatori economici in tutta la filiera ma il resto è prodotto dal consumatore finale. È dunque necessario agire da una parte sul fronte di educazione dei cittadini al valore del cibo e, dall'altra, facilitare la donazione da parte degli operatori economici. Noi abbiamo depositato qui in Senato un testo disegno di legge proprio per l'educazione al cibo e mi auguro che questo ramo del Parlamento possa al più presto farne partire il percorso parlamentare. stesso modo, nella legge di stabilità 2015 è stata inserita una norma che rende più conveniente per le imprese donare che buttare. Ci sono poi altri numeri che rappresentano la seconda faccia della medaglia e aumentano lo sconcerto. Sono i preoccupanti dati dell'ISTAT relativi all'aumento della povertà. Spreco alimentare e povertà sono un binomio inconciliabile, ma il metterli in relazione per ripristinare un equo riequilibrio non può avvenire secondo le regole del modello dell'economia di mercato che sono, di fatto, le stesse regole che hanno determinato tale squilibrio. Occorre un modello nuovo che, facendo leva anche su principi di eticità, consenta di rimettere in circolo ciò che non viene consumato, chiudendo il cerchio del ciclo di vita del prodotto secondo le regole dell'economia circolare, destinando le eccedenze a fini di solidarietà sociale. Bisogna sostenere la filiera della solidarietà, dal recupero dello spreco dei cittadini e degli operatori economici a nuovi consumatori finali. Nel Paese esistono già importanti risorse umane che, per vocazione e scelta personale, sono impegnate per la diffusione dei principi di giustizia sociale; si tratta del terzo settore e, restringendo il campo alla *mission* specifica, di associazioni che operano per il contrasto alla povertà e che hanno improntato il loro agire quotidiano secondo la logica della donazione, del

Questa è l'ambizione di questo provvedimento approvato alla Camera in un testo, che porta la firma di 217 deputati, risultante dall'unificazione di nove disegni di legge presentati dai partiti di maggioranza, dal M5S, da SEL e da FI. Un testo quindi largamente condiviso, che si è arricchito del contributo dato in audizione e con il confronto con tanti soggetti; condiviso al punto tale che molti di loro mi hanno pregato di preoccuparmi che questo testo non venisse modificato nel passaggio al Senato. Il testo mantiene la linea della legge n. 155 del 2003, detta «del buon samaritano», che, negli ultimi anni, ha regolamentato le donazioni e armonizza il quadro normativo per rendere agevole la donazione, attraverso semplificazioni e incentivi. Si riordina di fatto la materia delle cessioni ai fini di solidarietà sociale. Si affrontano i limiti più spigolosi di una burocrazia onerosa e di una normativa complessa, salvaguardando e garantendo la sicurezza degli alimenti e la tracciabilità dei prodotti. Veniamo ai contenuti del provvedimento, dei quali delineerò solo gli aspetti principali, vista l'ampiezza del provvedimento stesso, che si articola in tre capi, per complessivi 18 articoli. Il Capo I delinea, agli articoli 1 e 2, finalità e definizioni dei termini, indicando, tra le prime, la riduzione degli sprechi alimentari, farmaceutici e dei prodotti destinabili a fini di tipo sociale, per favorire il recupero e la donazione delle eccedenze e contribuire sia alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente, sia al raggiungimento degli obiettivi principali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, sia ad attività di ricerca e informazione dei consumatori. Il Capo II, comprendente gli articoli da 3 a 12, 3 a 12, contiene la parte più consistente del provvedimento, prevedendo misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale. L'articolo 3 detta, infatti, le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, da parte degli operatori del settore alimentare, alimentare, ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario. La cessione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano deve essere gratuita e rivolta prioritariamente a favore delle persone indigenti, mentre le altre eccedenze possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano e animale, le cui fasi di raccolta e ritiro saranno effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati. L'articolo 4 dispone sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari, consentita, a determinate condizioni, anche oltre il temine minimo di conservazione, per le quali è possibile l'ulteriore trasformazione nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza. Sono altresì previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico. L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita. L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca, stabilendo che l'autorità ne disponga la cessione gratuita a enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. Le disposizioni dell'articolo 7 possono essere lette in combinato disposto con l'articolo 13. Mentre infatti l'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti, l'articolo 13 amplia l'ambito della norma in base alla quale il soggetto che procede a distribuzioni gratuite di prodotti è equiparato al consumatore finale ai fini degli obblighi inerenti ai corretti stati summenzionati, con riferimento non solo agli alimenti, ma anche ai farmaci e a qualsiasi altro prodotto, sempre che essi siano distribuiti gratuitamente a fini di beneficenza. L'articolo 8 prevede l'integrazione delle funzioni e della composizione del tavolo permanente di coordinamento. L'articolo 9 contiene una serie di norme volte alla promozione e all'informazione in materia di riduzione degli sprechi. L'articolo 10 demanda al Ministero della salute la definizione di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità. L'articolo 11 provvede a rifinanziare con 2 milioni di euro per il 2016 il sopracitato Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituendo altresì un fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi. L'articolo 12 include la promozione di interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari tra le finalità del fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti. Dando per illustrato precedentemente l'articolo 13, continuo con l'articolo 14, che considera cessioni a titolo gratuito quelle di articoli ed accessori di abbigliamento usati. L'articolo 15 dispone in tema di medicinali inutilizzati, modificandone la disciplina sui sistemi dì raccolta e sull'eventuale successivo impiego. L'articolo 16 detta disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario, in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti. L'articolo 17 conferisce al Comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari, purché

Presidente, colleghi, la Commissione ha approvato diversi ordini del giorno, che rafforzano l'azione successiva del Governo, in particolare per la parte relativa agli sprechi farmaceutici. Mi avvio alla conclusione, ricordando che questa proposta di legge di iniziativa parlamentare raccoglie e riordina un percorso di norme degli ultimi vent'anni e crea una cornice omogenea: è ambiziosa perché si pone anche un obiettivo concreto che è quello di raddoppiare il recupero delle eccedenze. L'Italia vuol fare da traino per gli altri Paesi nella lotta agli sprechi alimentari, allargando sempre di più la platea dei donatori. Lo abbiamo reso possibile e continueremo a batterci per rendere sempre più semplici e naturali gli strumenti in grado di rendere la nostra società più giusta, più inclusiva e più equa.

la seduta è ripresa.

su un paio di aspetti che considererò meglio nel seguito. Ciò che però voglio segnalare è che siamo lontani dall'aspetto, che qualcuno invece ha ricordato, di somiglianza con la parabola del buon samaritano. Siamo molto più vicini a un'altra parabola del vangelo, quella di Lazzaro e del ricco Epulone. Ci troviamo, in pratica, a far parte di un sistema che spreca tanto perché è progettato male

lo sanno bene gli operatori del banco alimentare che si ritrovano sempre più richieste che disponibilità per accontentarli.

che reca in sé il progetto dello Stato del benessere e che si occupa della promozione dei singoli cittadini. Siamo molto più vicini alla carità cristiana, che è altra cosa, che toglie la fame, ma non restituisce l'orgoglio.

in questa, e della politica che il Partito Democratico e la maggioranza stanno ponendo in essere. dicevo, ogni anno la metà del cibo commestibile viene buttato via. una situazione in contrasto stridente con la fame di cui parlavo prima e, con i 4 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà. Nell'Italia che fa parte dei grandi,

viene fatto - è articolato, coordinato e complessivo se è vero, come è vero, che gli sprechi non si verificano in una fase specifica, ma in tutto il processo che dalla produzione

facilitano la cessione gratuita alle ONLUS che si occupano di assistenza, con una serie di precisazioni sugli aspetti fiscali della cessione. Definisce i requisiti perché dei beni siano considerati eccedenze impiegabili, tali da poter essere quindi avviate al recupero; istituisce un tavolo di coordinamento dove si possono formulare proposte per le politiche di filiera e condividere le buone pratiche.

Un punto importante di questa legge è il rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Tornando al discorso iniziale, l'espressione «distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti» a me sembra da testo ottocentesco. da testo ottocentesco. Vorrei che da questo punto di vista facessimo una riflessione importante. Siamo molto, molto distanti dallo Stato del benessere. D'altro canto, e ritorniamo ai limiti della politica, nell'articolato licenziato dalla Camera, che non è stato possibile emendare, non sono previsti elementi di obbligatorietà per accordi rivolti alla donazione delle eccedenze, accordi che dovrebbero essere resi obbligatori nei confronti della grande distribuzione, che ha un effetto di risucchio della ricchezza sia nei confronti dei consumatori sia nei confronti dei produttori (e lo sanno bene i produttori agricoli). Non è così dovunque. In Francia, per la mancata sottoscrizione di protocolli finalizzati alla distribuzione delle eccedenze si possono avere pene fine a 75.000 euro di multa o due anni di reclusione.

quest'Aula, limita la possibilità di incidere efficacemente nel senso che vogliamo, ossia nel senso della diffusione quanto meno di briciole di benessere. disegno di legge ha ancora aspetti positivi, se pensiamo al finanziamento della promozione di campagne di educazione alimentare nelle scuole, rivolte a ridurre gli sprechi. di vista mi preme segnalare un emendamento di Sinistra Italiana che trova la copertura necessaria per queste campagne di educazione alimentare nella soppressione delle vigenti agevolazioni fiscali sull'olio di palma, su cui l'IVA è ancora al 4 per cento e su cui l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riconosciuto la dannosità per la salute. Un'ultima cosa. Un altro aspetto che riteniamo debba essere tenuto in considerazione quando parliamo di donare farmaci la distribuzione e la somministrazione dei farmaci eccedenti dovrà avvenire attraverso l'impiego di personale dotato di adeguata formazione in campo sanitario; quindi il Governo deve provvedere a che questi aspetti sia attenzionati al massimo.

risultano ancora una volta intoccabili (quanto meno intoccati), e perché questo provvedimento appare come una pezza una pezza su una carenza di progettualità politica di ampio respiro, oppure su una politica di ampio respiro che considera la disuguaglianza come un tratto ineliminabile e, al massimo, da curare.

il disegno di legge che stiamo prendendo in considerazione persegue la finalità, sicuramente condivisibile, di limitare gli sprechi e incentivare la donazione e la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale, compresi i medicinali. Mi soffermerò in particolare sull'articolo 15 del disegno di legge in esame, che si occupa dell'utilizzo dei farmaci donati in favore delle organizzazioni senza fini di lucro e delle persone che si trovano in particolare condizione di bisogno, facendo prima una premessa e poi sottolineando alcuni aspetti, che meritano di essere posti all'attenzione dell'Assemblea e del Governo.

connesso contenente norme per la raccolta e la distribuzione di farmaci oggetto di donazione. In tale disegno di legge erano già indicati alcuni aspetti estremamente importanti, e sanità del Senato aveva svolto una serie di audizioni, compresa quella di un rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità, che ci avevano consentito di capire come meglio avrebbero potuto essere integrate le disposizioni presenti nel disegno di legge, in modo da garantire efficacia ai provvedimenti. Purtroppo il fatto che siano stati inseriti gli articoli, così come erano nel testo base, senza tener conto degli emendamenti sul quale avevamo svolto ampia discussione e su cui c'era un'ampia Commissione, ci impedisce di vedere, in questo momento, nel provvedimento che stiamo discutendo, alcuni elementi molto puntuali, che però renderebbero

In particolare avevamo studiato le modalità atte a favorire pratiche di donazioni appropriate per i beneficiari e i donatori donatori e, conformemente alle linee guida per la donazione di farmaci dell'Organizzazione mondiale della sanità, che sono state aggiornate recentemente, avevamo chiesto che fossero individuate delle modalità per proteggere i beneficiari da pratiche di donazione Ricordo che la letteratura scientifica riporta casi di donazione di farmaci contro l'obesità a Paesi del Centro Africa, che di norma hanno il problema opposto a quello dell'obesità. Quindi è importante che si

in modo più forte le responsabilità e il coinvolgimento dei destinatari nel processo di donazione, per garantire un adeguato coordinamento e un'efficace collaborazione tra donatore e destinatario in tutte le fasi del processo, nonché prevedere che le donazioni siano basate su bisogni espressi dei riceventi, nel rispetto delle politiche di tutela della salute e delle norme nazionali, anche attraverso il riferimento alla lista dei farmaci essenziali, che sono utili in condizioni di particolare bisogno, magari anche predisponendo delle linee guida nazionali per la donazione di farmaci. È difficile questi elementi possano essere inseriti in un provvedimento come quello che noi stiamo prendendo in considerazione oggi. Siccome l'impegno del Governo è quello di definire un decreto per dare attuazione al provvedimento,

credo che sia difficile trovare qualcuno in questa Assemblea che non condivida quantomeno la *ratio* del disegno di legge che stiamo per votare. Certamente è condivisibile la parte che riguarda gli alimenti, perché rimane impossibile concepire un mondo in cui ci sia chi spreca, mentre qualcun altro sta morendo di fame. Per renderci conto, diamo qualche numero della parte più povera del mondo: 795 milioni di persone che soffrono la fame, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo sprecato di cui 90 milioni solo in Europa: proprio nella nostra Europa, dove 16 milioni di persone si affidano alle organizzazioni caritatevoli per procurarsi cibo. E in questo campo si sono sviluppate, anche in Italia, procedure ormai collaudate per la raccolta e la distribuzione di derrate alimentari scadute, ma ancora buone e utilizzabili, che danno risultati tangibili ogni giorno, per consentire a tantissime persone di mangiare del cibo ancora valido senza rischi per la salute. Ma questo disegno di legge si occupa anche di un altro aspetto, altrettanto importante perché attiene all'uso dei medicinali. Per questo vorrei immediatamente evidenziare che il farmaco oggetto di donazione non ha le stesse caratteristiche del cibo. Le peculiarità del farmaco stanno nelle proprietà curative e profilattiche delle malattie dell'uomo. Per mezzo del farmaco si attua una terapia a difesa della salute. Devo quindi ricordare, ai fini del Resoconto, che l'immissione in commercio di medicinali prevede un *iter* assai puntuale che ne disciplina la produzione, l'autorizzazione, la messa in commercio, la distribuzione, l'informazione medico-scientifica e infine anche la farmacovigilanza, cioè il controllo dopo la vendita.

Quindi, ancor più e ancora meglio di qualsiasi approccio si possa tenere nei confronti dei generi alimentari, che è giusto recuperare finché non evidenzino i minimi segni di alterazioni, per i farmaci bisogna usare certamente maggiore cautela proprio per evitare possibili rischi sulla salute dell'uomo. In questo senso, nel caso della donazione del medicinale, entra in gioco la necessità di garantire la scurezza del paziente. E come si può garantire davvero questa sicurezza? La sicurezza del paziente la si garantisce tutelando chi è oggetto di una donazione, come la legge italiana tutela chiunque acquisti un farmaco. Nell'articolo 15, infatti, non si menziona il garante della dispensazione, cioè il farmacista, che è la garanzia che la norma italiana prevede per la sicurezza del paziente all'atto della dispensazione di un farmaco, sia esso da banco o sottoposto a prescrizione medica. Infatti, quando abbiamo di fronte una donazione abbiamo i due casi classici. Quello di un farmaco da banco, del quale farmacista è il garante della appropriatezza dell'assunzione del farmaco, ma anche la garanzia per il cittadino di avere tutte le informazioni necessarie per assumerli in sicurezza. Oppure, abbiamo farmaci con obbligo di presentazione medica e, quindi, ancora di più la necessità di qualcuno che possa filtrare la richiesta del cittadino e che possa quindi dare una risposta reale alla sua esigenza di malattia.

potendosi avvalere della consulenza qualificata del farmacista e di chi, invece, non ha i soldi ma necessita dello stesso consiglio, per una scelta che ha ricadute ovvie sulla sua salute. Non possiamo pensare che, siccome si tratta di un dono, il controllo sull'appropriatezza dell'utilizzo non sia importante. Dirò di più: senza l'introduzione di una figura professionalmente qualificata come il farmacista all'atto della dispensazione, chi potrà innanzitutto valutare se davvero il rimedio è giusto per la persona che ne ha bisogno? Ma di più, chi potrà consigliare la posologia, assicurarsi che sia quella giusta e sapere quando prendere questo farmaco, se prima o dopo il pasto, e quante volte al giorno? E come si potrà dare un consiglio sulla conservazione? Questo è il grave *vulnus* dell'articolo 15: non è prevista una presenza, che è garanzia della sicurezza dell'assunzione di un farmaco. Per questo, secondo me, quello che manca nell'articolo 15 è proprio l'introduzione obbligatoria della presenza del professionista come imprescindibile strumento per garantire la sicurezza del paziente.

Concludendo, le donazioni di farmaci devono seguire una procedura che comporti una rigorosa verifica. Per questo ritengo fondamentale, per i motivi che ho illustrato, che la specifica disciplina delegata dall'articolo 15 al Ministro della salute e relativa alla raccolta di medicinali inutilizzati, alla donazione e all'impiego dei medesimi, debba farsi carico di alcune prescrizioni ulteriori rispetto agli altri beni oggetto di donazione. Dalla qualità del processo distributivo e sino alla dispensazione finale deve essere messa in primo piano la tutela della salute del cittadino. anche per i farmaci raccolti per queste finalità è necessario fornire tutte, ma proprio tutte, le medesime garanzie fornite attraverso la dispensazione del farmaco in farmacia.

di cui abbiamo esaminato gli emendamenti. L'articolo 40 del nostro Regolamento prevede che i pareri della 5a Commissione siano considerati obbligatori al punto che tutte le Commissioni sono tenute a inviare il testo base e i relativi emendamenti che ad esso sono attribuiti perché la 5a Commissione possa possa esprimere un parere che diventa addirittura ostativo rispetto alla sede redigente o deliberante e determina il trasferimento in Aula del provvedimento. Noi abbiamo proceduto alla votazione degli emendamenti in questo momento scopriamo che la Commissione bilancio non aveva espresso questi pareri. Io so che in passato in sede referente si è superato questo problema e comunque si è andati

del decreto-legge, cosa che non credo riguardi il decreto-legge in oggetto, perché abbiamo ancora la giornata di domani e di dopodomani per poterlo esaminare e credo che al massimo nella giornata odierna o in 5a Commissione avrebbe potuto e avuto modo di potersi esprimere. Ricordo che numerose volte ho trovato già in Commissione in sede referente il parere contrario ai sensi dell'articolo 81

Signora Presidente, lo spreco alimentare di cui parliamo oggi è divenuta questione impellente nel dibattito europeo e mondiale. È opportuno e necessario che, dopo la Francia, anche l'Italia si doti di un testo di legge con queste caratteristiche e questa natura anche per una lotta all'inquinamento ambientale e alle diseguaglianze tra le diverse aree del pianeta,

e non è più possibile non provare a fornire soluzioni concrete per sconfiggerlo. Era uno degli impegni che ci eravamo assunti con il ministro Martina qui presente al Protocollo di Milano, che poi è diventato il nostro manifesto: 868 milioni di persone soffrono la fame nel mondo, un miliardo e mezzo però sono gli obesi; ogni anno muoiono 36 milioni di persone per fame mentre 29 milioni muoiono per eccesso di cibo. L'umanità butta un terzo della sua produzione alimentare, quattro volte quello che basterebbe per sfamare quegli 868 milioni di persone che non ce la fanno. In più, un terzo dei raccolti è impiegato per biocarburanti e mangimi e la domanda sta salendo. Attualmente consumiamo una quantità di risorse che supera di una volta e mezzo quanto la Terra possa obiettivamente produrre in un anno; se continuiamo a procedere di questo passo avremo bisogno di tre pianeti che proprio non ci sono. Stando alle proiezioni del consumo futuro, quello intensivo soprattutto metterebbe in ginocchio gli ecosistemi esistenti, oltre a rendere i nostri prodotti, quelli che arrivano sulle nostre tavole, assolutamente privi del valore qualitativo di cui abbiamo bisogno.

Perdite e sprechi si verificano ad ogni stadio della filiera alimentare ed è stato opportuno per tale ragione mettere in campo una serie di azioni che si sono articolate nelle

di lasciare da parte, ciascuno di noi, come diceva poc'anzi anche la collega Dirindin, le proprie volontà di inserimento di ulteriori elementi valutativi, al fine di permettere il passaggio finale di questo importante progetto, affinché l'Italia faccia la sua parte fin da subito.

Va sottolineato - e questo mi compete come componente della Commissione ambiente e come persona informata sui fatti - che ogni grammo di cibo sprecato diventa anche un grammo di rifiuto da smaltire. Il costo ambientale, quindi, si accresce e diventa più pesante. Sarebbe forse arduo quantificare il danno ambientale ed economico che viene causato quando ancora il cibo non è entrato in contatto col cliente finale.

pari al fabbisogno annuo di più di 8 milioni di italiani. Allo stesso modo, vengono prodotti 24,5 milioni di tonnellate di biossido di carbonio, un quantitativo inquinante pesante

uno a mia prima firma - che introducono un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di merci che distributori e produttori smaltiscono in maniera corretta, dandola direttamente alle associazioni che si occupano di indigenti o di aventi bisogno; definisce come sia indispensabile - lo abbiamo scritto nel testo - che si provveda fin d'ora a creare una cultura alimentare anche nelle scuole. La dico così: dopo i nativi digitali, noi vorremmo che i nostri figli, possibilmente già da ora, diventassero nativi ambientali, cioè si rendessero pienamente conto delle conseguenze di ogni gesto e di ogni scelta

nei prossimi anni la produzione alimentate del 60-70 per cento, per nutrire una popolazione sempre crescente, dall'altro si spreca nel mondo oltre un terzo del cibo prodotto, di cui l'80 per cento sarebbe ancora consumabile, cioè utilizzabile ai fini della nutrizione. Lo spreco alimentare è tanto più illogico quanto più aumentano la produzione di rifiuti e la crisi ambientale, nonché l'impoverimento e la denutrizione (oltre 1 miliardo di persone attualmente sono denutrite). Autorevoli fonti affermano che, se fosse possibile recuperare gli sprechi alimentari, si riuscirebbero a sfamare circa 2 miliardi di persone miliardi di persone al mondo. Gli sprechi riguardano tutti i passaggi che portano gli alimenti dal campo alla tavola e colpiscono indistintamente tutti i Paesi. L'Unione europea, con 180 chilogrammi *pro capite*, e l'Italia, con 149 chilogrammi *pro capite*, risultano sopra la media dei Paesi sviluppati nella classifica dei Paesi spreconi. Nel nostro Paese gli sprechi a livello domestico sono i più rilevanti, il 42 per cento del totale, e costano oltre 25 euro al mese a famiglia. Possiamo constatare che un cibo che non nutre nessuno non solo è inutile, ma è anche dannoso. Con il cibo buttato vengono infatti sprecati anche la terra, l'acqua e i fertilizzanti (senza contare le emissioni di gas serra) che sono stati necessari per la sua produzione; l'ambiente è stato quindi inquinato, sfruttato o alterato invano. Ed è stato sprecato anche il lavoro umano, che, in quei casi non rari in cui il lavoro è sfruttamento di manodopera, assume le sembianze della beffa agroalimentare, perché quel lavoro non è servito a sfamare. Combattere lo spreco alimentare e le sue conseguenze ambientali è una delle missioni caratterizzanti il terzo millennio. In molti casi, sono sufficienti semplici azioni da parte di singoli cittadini (produttori, rivenditori, ristoratori, aziende della trasformazione) per contribuire a raggiungere la sicurezza alimentare e una migliore sostenibilità ambientale. L'articolo 1 spiega nello specifico le finalità del disegno di legge: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti (ad esempio (ad esempio l'abbigliamento) a fini di solidarietà sociale; ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riuso e il riciclo, contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della legge. Attualmente le imprese, i ristoratori e i supermercati della grande distribuzione organizzata che vogliono donare le eccedenze devono presentare una dichiarazione cinque giorni prima. Con la nuova legge basterà invece una dichiarazione di riepilogo a fine mese, che garantisca la tracciabilità di quello che si è dato. Dal documento di trasporto e dagli scontrini potrà essere scaricata l'IVA e la legge prevede un possibile sconto sulla tassa dei rifiuti, proporzionale alla quantità di cibo donato. Gli operatori del settore alimentare potranno cedere gratuitamente le eccedenze, se vorranno farlo, alle associazioni di di volontariato, che le ritireranno direttamente e le destineranno «a favore di persone indigenti». L'articolo 16 del testo unificato allarga la platea degli operatori che potranno ritirare le eccedenze, prima riservata solo alle ONLUS,

nei ristoranti l'uso di contenitori per portarsi a casa gli avanzi. La legge dice anche che le Regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Stiamo parlando della *family La legge interviene infine sui consumatori. Gli sprechi alimentari riguardano infatti non soltanto i produttori, i distributori, e tutti i dispensatori di cibo al pubblico, ma anche i consumatori che producono il 43 per cento degli sprechi stessi. Per questo la proposta chiede una vasta sensibilizzazione sul tema in modo da rendere più consapevoli del problema tutte le parti in causa. La RAI, con i suoi canali televisivi televisivi e radiofonici, generalisti e tematici, in quanto ente pubblico, dovrà assicurare un adeguato numero di ore dedicate all'argomento. La proposta di legge punta dunque sugli incentivi, sulla semplificazione burocratica e sulla creazione di un sistema che oltre le singole iniziative risolva il problema, ma di fatto non prevede alcun obbligo. L'analoga legge francese prevede invece sanzioni. Inoltre, il disegno di legge non interviene per nulla nella prevenzione, sul contrasto alla sovrapproduzione di cibo, sulla pressione che l'industria alimentare esercita sulle nostre scelte, attraverso una pubblicità incontrollata e non regolata, che crea veri e propri bisogni indotti, convincendoci che abbiamo bisogno di più più cibo di quello che, in realtà, ci necessita, e convincendoci a comprare una quantità sempre maggiore di cibo e di sempre più scarsa qualità. Poi, se il cibo si consuma o si butta, in realtà, poco importa, l'importante è che si venda. Lo spreco alimentare, infatti, non è solo il cibo che scade sugli scaffali e che viene gettato dai supermercati. Per combattere lo spreco alimentare, è importante ridurre, appunto, questi 2,5 milioni di tonnellate annue di derrate che buttiamo nelle nostre case. Queste derrate alimentari sono arrivate nei nostri domicili perché, magari, siamo stati condizionati all'acquisto

e sempre di fretta può essere anche una patologia; potevamo migliorane il testo, ma questa maggioranza evidentemente non ha voluto far proprio ciò che Plutarco ci ha insegnato, ovvero che la facilità e la velocità nel fare una cosa non danno al lavoro durevole solidità, né la precisione della bellezza. C'è uno *slogan* che può essere fatto proprio dalla comunità nazionale nel Paese che vorrebbe perseguire l'ideale della bellezza: bello, buono e ben fatto caratterizzano infatti il *made in Italy*. Anche il vergognoso prezzo del grano coltivato nei nostri campi, esempio per tutti, può rientrare nella *plèiade* dei prodotti cui occorre prestare un'attenzione etica, morale, una dignità civica ed educativa nazionale. Che il cibo si consumi o si butti in realtà non importa, che le persone si ammalino in realtà non importa, l'importante è che cresca il PIL, il prodotto interno lordo. L'importante è che il disegno di legge non venga appesantito. L'importante è che il Governo possa fare uno dei soliti *tweet*

leggevo delle agenzie che riguardano la Turchia, con Erdogan che vuole inserire la pena di morte e se la prende con l'Italia perché c'è un'indagine in corso nei confronti del figlio per riciclaggio, l'ambasciatore russo definisce illegittime le azioni di bombardamento degli Stati Uniti sulle postazioni dell'ISIS. Noi, invece, siamo qui a parlare dello spreco alimentare. Cosa è fuori posto? Noi o il mondo che sta fuori?

porti ad essere più distratti rispetto a queste circostanze, costituisce invece un momento di progresso civile. Tutti noi abbiamo più o meno ereditato dalle nostre famiglie o dalle nostre

se solo riscoperte o riconsiderate, ci portano a valutare come l'esperienza e la saggezza di un tempo facevano sì che non si sprecasse nulla. Esistono oggi piatti in tutte le tradizioni regionali italiane che nascono dal riuso degli alimenti,

Secondo una tradizione, diffusa soprattutto nel Nord Italia, del maiale, per esempio, non si butta via nulla. Il Ministro, che viene dall'area prealpina, sa benissimo di cosa parlo. Stiamo parlando però di un tempo che appare abbondantemente superato e, infatti, in un *fast food*, trascorsi cinque minuti, se le patate si raffreddano vengono gettate nella spazzatura. Queste sono due situazioni che stanno agli antipodi. La globalizzazione del McDonald's non ci fa più ricchi in questo senso. Dimenticare e perdere questa considerazione nei confronti dell'alimento è un impoverimento per tutti noi. Se oggi abbiamo qualche soldo e qualche ricchezza in più, che ci consente di far arrivare sulle nostre tavole cibo in abbondanza, dobbiamo ricordarci sempre del valore alimentare e della fatica che sta dietro la produzione. Questo provvedimento di legge ha in se stesso un'importanza che definirei etica. Viene dopo provvedimenti che, nel nostro Paese, hanno già percorso la strada del combattere lo spreco di cibo. Penso alla cosiddetta legge del buon samaritano,

di non cadere nella tentazione di essere universali nell'affrontare una questione. È infatti meglio essere precisi e puntuali, svolgendo bene un compito, piuttosto che inserire più argomenti e temi che rischiano poi di creare confusioni o difficoltà attuative,

dei cittadini che debbono essere tenuti in seria considerazione. Un pezzo di pane secco è cosa ben differente da un farmaco ancora integro, ma distribuito. Bisogna fare attenzione a non mescolare troppi argomenti, così rendendo un cattivo

in merito al pesce azzurro, che viene pescato nei nostri mari e che non viene importato, ma di cui sappiamo che solamente una minima parte

Questo è un errore. Nella tradizione sappiamo che l'aguglia, la leccia, l'alice, la costardella, il lanzardo, il pesce sciabola, la sardina, il sugarello e lo sgombro (potremmo elencarne altri) sono pescati nei nostri mari

Non si potrà arrivare seriamente a una limitazione degli sprechi alimentari se non si sviluppa, o - tornando a - tornando a quanto dicevo prima - non si recupera una cultura del valore del cibo che abbiamo nel piatto: ciò che viene raccolto dall'agricoltore, ciò che viene pescato dal pescatore e ciò che viene allevato dall'allevatore. Se non si riprende a sviluppare una considerazione del valore del prodotto e dell'alimento avremo sempre una battaglia tra uno sgravio fiscale e un'attenzione contributiva, ma - ahimè - temo destinata alla frustrazione. Il rapporto fondamentale da recuperare è quindi quello tra famiglia, scuola e società è importante - indirizzo ancora un appello al Governo - sostenere e finanziare seriamente politiche di sviluppo della cultura e della considerazione a partire dai più giovani riguardo al recupero degli alimenti.

Sì, ma è soprattutto un'eredità che ci viene dal passato; per chi è a conoscenza di quella che è stata la nostra miseria, essere oggi seri nel consumo alimentare significa portare rispetto a chi è venuto prima di noi e alle generazioni che hanno fatto fatica prima di noi.

*(Misto)*. Signora Presidente, gentili colleghi, sono contenta che oggi siamo giunti a discutere una proposta legislativa che affronta la problematica degli sprechi, in particolare di quelli alimentari. Tra le molteplici e condivisibili finalità del provvedimento, accolgo con favore l'intento di contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori, con particolare riferimento alle giovani generazioni. a cuore questa delicata tematica dalle molteplici implicazioni: la lotta agli sprechi è stata infatti oggetto di due disegni di legge da me presentati. Penso che siamo tutti consapevoli del fatto che, in un contesto globale di pesanti diseguaglianze economiche e sociali, risulti inaccettabile il perdurare di situazioni endemiche di sprechi alimentari. Ricordo che a suo tempo mi colpì molto il paradosso che emerge dalla lettura dei dati della FAO: circa 805 milioni di persone nel mondo soffrono la fame ogni giorno, mentre 1,5 miliardi risultano obese. Il fenomeno dello spreco alimentare, a livello globale, risulta quindi degno della massima attenzione. Cito brevemente qualche altro dato solo per dare un'idea di massima della serietà dello scenario che abbiamo di fronte. Il volume globale di spreco alimentare sia aggira attorno a 1,6 miliardi di tonnellate, e di questi la parte di spreco di cibo commestibile ammonterebbe a 1,3 miliardi di tonnellate. Per quanto concerne l'Europa, secondo studi eseguiti su incarico della Commissione europea, circa 100 milioni di tonnellate di cibo vanno sprecate all'interno dell'Unione e in assenza di misure, quindi di cambiamenti significativi, si potrebbe arrivare a 120 milioni di tonnellate nel 2020. Occorre poi tenere presente un altro effetto della problematica in esame. Lo spreco alimentare, oltre a costituire una rilevante questione etica e a provocare danni a livello economico, rappresenta anche un serio pericolo in termini ambientali, visto che depaupera in maniera significativa il bacino delle limitate risorse del pianeta. Si pensi solo al fatto che il volume di acqua utilizzata annualmente per produrre cibo che poi va sprecato è equivalente al flusso annuale del Volga o a tre volte il volume del lago di Ginevra. Le conseguenze economiche dirette derivanti dagli sprechi alimentari sono stimate intorno ai 750 miliardi di dollari all'anno. Per quanto concerne l'Italia, secondo il rapporto 2014 Waste Watcher-knowledge for Expo, ogni anno 5 milioni di tonnellate di prodotti alimentari finiscono nella spazzatura. Si parla di una cifra attorno agli 8 miliardi di Europa, pari a mezzo punto di PIL. Quanto descritto non può lasciare indifferenti. Alla luce di dati sempre più allarmanti, ricordo che già nel 2012 il Parlamento europeo, mediante la risoluzione 2011/2175 indirizzata alla Commissione europea, esortava all'adozione di misure concrete per porre fine, entro il 2025, allo spreco di cibo all'interno del territorio dell'Unione. Penso quindi che questo sia un obiettivo da perseguire con la massima serietà e in questo senso tutti i Parlamenti dell'Unione condividono una responsabilità. Pertanto, la proposta legislativa che oggi ci accingiamo a votare rappresenta, a mio avviso, un primo passo avanti nella direzione di una sempre maggiore consapevolezza e volontà di arginare

all'interno del territorio nazionale. Spero quindi che riceveranno sostegno gli emendamenti che ho presentato sul tema e che prevedono, per l'appunto, tale obbligo. Mi auguro, dunque, che questo sia solo l'inizio di un percorso virtuoso, che veda il coinvolgimento sinergico di istituzioni e società.

il provvedimento che discutiamo oggi è tanto utile quanto poco costoso, non solo economicamente, ma anche dal punto di vista dell'introduzione di nuove regole o divieti. L'idea che sta alla base, infatti, è quella di recuperare e donare le eccedenze alimentari o di altri prodotti, affinché possano essere utili a persone che ne hanno bisogno. Facendo ciò contribuiremo, oltre che al rafforzamento del sentimento di solidarietà sociale, anche alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente, che derivano dal ciclo di produzione dei beni. Questo è ancora più vero il disegno di legge in esame introduce politiche volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo, anche incoraggiando le attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini. Gli articoli 3 e 4 del testo delineano il sistema grazie al quale prodotti alimentari e agricoli, ancora commestibili, ma scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche, o perché vicini alla scadenza, saranno destinati a persone indigenti. Il tramite sarà rappresentato da tutti quegli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. Da parte loro, gli operatori del settore alimentare, che effettuano le cessioni a titolo rigorosamente gratuito,

dei comportamenti virtuosi di riduzione degli sprechi, disponendo che la RAI, attraverso le proprie trasmissioni televisive e radiofoniche, diffonda messaggi di informazione e sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi alimentari ed energetici. Toccherà al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il compito di promuovere campagne nazionali di comunicazione, per diffondere modelli di consumo e di acquisto solidali e sostenibili, oltre a piani di recupero e redistribuzione per fini di beneficenza. L'articolo 11 prevede il finanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, con 2 milioni di euro per il 2016. Inoltre, si istituisce un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro annuo fino al 2018, per finanziare progetti innovativi, che favoriscano la limitazione degli sprechi e la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Viene incrementata anche la capacità finanziaria del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, con ulteriori 2 milioni di euro. Come accennato all'inizio, però, il disegno di legge non trascura il riuso di beni e prodotti ulteriori rispetto alle derrate alimentari. È importante ricordare, infatti, anche le disposizioni dell'articolo 14, dedicate alle cessioni a titolo gratuito di articoli ed accessori di abbigliamento effettuati direttamente Oltre ai beni alimentari e di abbigliamento, si interviene con l'articolo 15 anche sui sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati, semplificando le procedure burocratiche per l'elaborazione per l'elaborazione delle norme di settore e circoscrivendo l'ambito di azione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Per garantire la sicurezza per la salute di tali medicinali, viene introdotto il requisito delle confezioni integre e viene prevista l'esclusione di alcune categorie di farmaci, come ad esempio medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, o contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Vorrei ricordare, in conclusione, come la norma dell'articolo 17, in modo condivisibile e virtuoso consente ai comuni di ridurre la tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche (la TARI) per quelle attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che ne donano una parte agli indigenti o per l'alimentazione degli animali. Un provvedimento, quindi, di avanzata civiltà che consente l'uso efficiente di qualsiasi risorsa, sia essa alimentare o materiale, al fine di aiutare il prossimo più bisognoso. Un provvedimento, e lo sottolineo, che rafforza ancora di più la posizione dell'Italia in prima linea nell'ambito della tutela dei diritti essenziali delle persone. Nell'auspicare l'approvazione da parte dell'Assemblea del

Signora Presidente, vorrei segnalare in premessa che l'andazzo del Governo di prendere provvedimenti in studio nelle varie Commissioni ed inserirli nei decreti è, ad oggi, anche appannaggio della Camera. Infatti, in questo provvedimento se ne è ripreso un altro analizzato dalla Commissione sanità sulla distribuzione dei farmaci, l'Atto Senato 1092 e seguenti, sviscerato e già emendato, pronto per essere licenziato, che viene inserito in maniera incompleta e imparziale, delegando al Governo, con apposito decreto, la risoluzione di quelle criticità già risolte dalla Commissione. Ma la necessità di licenziare la legge ne ha impedito l'implementazione e, pertanto, sono state fatte integrazioni con alcuni Il provvedimento che andiamo ad analizzare si concentra più sulla gestione degli sprechi, che sull'evitarne la formazione. La dimostrazione di questo enunciato sta nel comma 3 dell'articolo 4, dove vengono considerati eccedenza alimentare «i prodotti «i prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti non essendo stati venduti o somministrati entro le 24 ore successive alla produzione». I nostri nonni facevano un pane che manteneva le caratteristiche di consistenza per una settimana. Noi lo consideriamo rifiuto dopo 24 ore. È evidente che c'è un approccio produttivo sbagliato e su questo la legge non si esprime se non con vaghi enunciati privi di concretezza, come all'articolo 1, comma 1, che introduce «la finalità di ridurre gli sprechi della fasi di produzione», ma non dà alcuna indicazione.

Invece, si lascia al cittadino la scelta di optare per l'acquisto di quei prodotti, che hanno un costo economico lievemente superiore, ma sono sostenibili e rispondono ai requisiti di eticità. Questo provvedimento regolamenta le varie fasi della raccolta e distribuzione delle eccedenze, individua anche fondi (modesti e su vari capitoli, forse troppi), dà agevolazioni IVA, riduce la tariffa relativa alla tassa dei rifiuti e nel contempo aiuta persone in difficoltà. altre criticità riscontrate solo come elemento di riflessione e di analisi. Ad esempio, la definizione di «soggetti cessionari» ovvero i soggetti che possono attuare la cessione gratuita agli indigenti. Il testo approvato, in luogo delle attuali ONLUS, amplia in maniera indefinita la platea, includendovi l'intero terzo settore e non escludendo, ad esempio, le imprese sociali, che tendenzialmente operano come operatori nel mercato e non dovrebbero praticare «attività di beneficenza». è costituito dall'introduzione della tracciabilità delle cessioni, il rispetto del principio della rotazione, della trasparenza e dell'evidenza pubblica. Ciò al fine di evitare che tali cessioni avvengano esclusivamente a favore dei medesimi enti e sfavorire quindi possibili traffici o accordi illeciti o non trasparenti. In tal senso si può pensare d'introdurre la possibilità che sui siti istituzionali dei Comuni siano previste sezioni dedicate all'economia circolare. Inoltre, al fine di rendere efficace l'obiettivo della legge, è importante che si realizzi anche un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella filiera agroalimentare e che in tal senso siano definite a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti, con indicazione dei soggetti della filiera obbligati obbligati a fornire le informazioni delle cessioni. Un'altra criticità è connessa al fondo presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 11). La proposta in esame tratta in maniera congiunta il citato fondo che, diversamente dalle finalità del presente disegno di legge, non è mirato alla riduzione dello spreco alimentare, ma alla distribuzione di derrate

Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi senatori: «La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti». Con queste parole inizia il disegno di legge che stiamo esaminando, l'Atto Senato 2290, che reca il titolo «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi». Con queste premesse, chi può essere contrario alle finalità ed allo spirito di questo disegno di legge? Vorrei anzi sottolineare come Forza Italia sia sempre stata a favore della lotta allo spreco, ricordando che nel 2003 il Governo Berlusconi varò la legge detta del buon samaritano che, tra le prime in Europa, consentì in Italia la donazione di alimenti per i più bisognosi. Oggi, oltre alla possibilità di donare le derrate alimentari che risultano in eccedenza, si aggiungono sia la possibilità di donare farmaci non utilizzati (ovviamente con rigide regole per la tutela della salute), sia una sostanziale semplificazione per la donazione di abiti e di accessori di abbigliamento. Voi pensate quindi che tutto vada bene, ma non è proprio Onorevoli colleghi, stiamo vivendo una crisi che ha avuto inizio nell'ormai lontano 2007 e che è esplosa a livello mondiale nel 2008: otto anni in cui la crisi è stata dura, durissima, e ha portato anche in Europa la recessione, l'aumento della disoccupazione, la povertà ed addirittura la fame, spettri che credevamo di esserci lasciati definitivamente alle spalle. L'ISTAT ci dice che nel 2015 ancora 1.582.000 famiglie italiane vivono in condizioni di povertà assoluta, pari a più di 4,5 milioni di persone e questo è il dato peggiore dal 2005. Chi sostiene che la crisi è passata deve fare i conti con questi numeri. Questo è il quadro reale della situazione ed è in questo contesto, tutt'ora irrisolto, che dobbiamo valutare l'efficacia di questo provvedimento. Mi viene quindi di dire che è troppo poco. Mentre è apprezzabile, infatti, l'attenzione normativa, la voglia di aiutare chi si adoperi per il bene dei più sfortunati, in piena sintonia con il concetto di sussidiarietà e di equivalenza dell'iniziativa privata con quella pubblica, in discussione non c'è traccia di quella rivoluzione culturale, di quel cambio di passo necessari perché si affronti alla radice lo scandalo dello spreco alimentare che, come dice la FAO, costa ogni anno al mondo 1.000 miliardi di euro. Avremmo dovuto fare di più, soprattutto con l'aumento delle coperture economiche, perché è nell'aiutare chi ha bisogno che si misura il grado di civiltà di un Paese. Forza Italia ha proposto, sia alla Camera che al Senato, un aumento delle risorse a disposizione. Si potevano, per esempio, creare maggiori incentivi fiscali per le società che volessero donare, con detraibilità fiscali adeguate. Si sarebbero potute trovare soluzioni più efficaci della sola possibilità (lasciata alla buona volontà e all'attenzione dei Comuni) di applicare sconti sulla TARI per le società che donano alimenti o farmaci. C'è un altro elemento di criticità che vorrei sottolineare. Tutto il disegno di legge è impostato sul concetto di donazione spontanea. Mi domando se non sarebbe stato meglio affrontare il tema dello spreco in materia più radicale, trovando la maniera di obbligare in qualche modo alcuni soggetti (penso per esempio alla grande distribuzione, alle catene di *fast food*) a donare le rimanenze, soprattutto quelle alimentari. Sarebbe stato un segnale forte e preciso, soprattutto in questi momenti di difficoltà, e avrebbe aiutato il Paese a raggiungere l'obiettivo «fame zero» entro il 2030, così come stabilito dalla Carta di Milano e dai nuovi obiettivi del Millennio dell'ONU. Proprio per supportare questi obiettivi, avevamo proposto, con un nostro emendamento, di creare a Milano, sede dell'Expo 2015, l'osservatorio che dovrebbe contribuire a facilitare questo percorso. Avevamo sperato che, dopo il passaggio alla Camera, il Senato avrebbe potuto migliorare il provvedimento con emendamenti mirati, ma ancora una volta, come sta succedendo troppo spesso ultimamente, ci è stata vietata la possibilità di intervenire. Ciò detto, si deve anche riconoscere che il provvedimento presenta aspetti positivi, come per esempio la possibilità di donare confezioni di cibo anche oltre il termine minimo di conservazione, o quella di donare i materiali alimentari confiscati dalle autorità agli operatori pubblici o privati che perseguono, senza fini di lucro, finalità civiche o solidaristiche. È una buona cosa, inoltre, che si prevedano campagne di comunicazione di RAI, Ministero delle politiche agricole,

cosa che è certamente alla nostra portata, dobbiamo modificare le nostre abitudini, comprendendo che è un dovere morale smettere di buttare cibo ancora commestibile quando tanti nostri compatrioti hanno difficoltà a mangiare due volte al giorno. Credo, in conclusione, che questo sia uno dei casi in cui valga il concetto che è meglio poco che niente, perché il poco che è qui previsto sarà comunque un aiuto concreto ai milioni di persone che in Italia vivono in stato di indigenza.

signor Ministro, signor Vice Ministro, cari colleghi, ho sentito emergere da tutti gli interventi una generale convergenza e una positività generalizzata, che non è cosa da poco. Infatti, questo disegno di legge persegue finalità, oggi più che mai necessarie, di riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari. (è l'aspetto che vorrei sottolineare come elemento assolutamente positivo del provvedimento) deve partire, a mio parere, dal mondo della formazione e della scuola, come peraltro qualcuno ha accennato. Andrebbe valorizzato in tal senso il ruolo degli istituti scolastici in generale e, in particolare, quello degli istituti tecnici agrari e professionali con annesse aziende, il mondo dell'istruzione e della formazione professionale (alberghieri, indirizzi di cuochi, camerieri). È assolutamente importante valorizzare questo elemento attraverso i vari indirizzi. Il processo educativo dovrebbe coinvolgere tutto il mondo della scuola, incluse le mense scolastiche, come ho avuto modo di rilevare di rilevare in 7a Commissione, che ha ampiamente discusso su questo provvedimento. Contribuire ad azioni positive per limitare gli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il tempo di vita dei prodotti significa contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Ma significa anche di più. Il potenziale del riuso per i viventi implica una sfera etica, una serie di valori da cui non possiamo prescindere: quelli della solidarietà sociale, dell'attenzione alle fasce deboli, del rispetto dell'ambiente. Sappiamo che i beni ambientali non sono inesauribili, per cui la cultura del non spreco deve sostituirsi all'incultura, alla banalità dell'usa e getta, un usa e getta a cui la comunità educante ha guardato nel passato forse con troppa superficialità, senza linee educative forti di contrasto, a volte persino abdicando ad un ruolo fondamentale. Ed è ai giovani che va trasmessa una formazione culturale diversa, una cultura della donazione e un'etica della responsabilità e della consapevolezza dell'impatto sull'ambiente di ogni nostro gesto. Ciascuna azione, ciascun bene consumato lascia un'impronta ecologica più o meno sostenibile. Sta in noi saper amministrare le nostre impronte, non consumare in eccesso o consumare senza errori eccessivi, attraverso un riutilizzo positivo che non intacchi in modo irreversibile le risorse da destinare alle future generazioni. Sono questi il senso, la *ratio* e la filosofia La Carta di Milano, che in molti abbiamo sottoscritto e condiviso, è richiamata in questo disegno di legge, quando fa riferimento al diritto di tutti ad una quantità sufficiente di cibo, sano e nutriente, che soddisfi le necessità alimentari personali; quando richiama alla consapevolezza una delle maggiori sfide dell'umanità sarà quella di nutrire una popolazione in costante crescita - come ha detto qualcuno poc'anzi - senza danneggiare l'ambiente; quando richiama gli impegni alla cura del cibo di cui ci nutriamo. legge prevede un'attività di corretta informazione e sensibilizzazione dei consumatori, che deve coinvolgere i *media*, il servizio pubblico radiotelevisivo, le istituzioni, il mondo della formazione e della ricerca, per indurre comportamenti improntati a criteri di solidarietà e sostenibilità. Esso prevede inoltre, per chi attui la cessione gratuita degli alimenti al fine di solidarietà sociale, procedure semplificate che incoraggino produttori, distributori e trasformatori. Questo è previsto dal Capo II, dove il disegno di legge invita a dare priorità nelle donazioni agli indigenti, ferma restando la piena garanzia sull'integrità dell'imballaggio primario e delle idonee condizioni di conservazione.

dando ai Comuni la facoltà di applicare alle imprese, alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono tali beni alimentari agli indigenti, un coefficiente di riduzione della tariffa di asporto rifiuti, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. È davvero un'importante opportunità, che auspico i sindaci vogliano cogliere convintamente, poiché i benefici ricadono sulla collettività. Cito l'articolo 7, che coinvolge il mondo degli enti pubblici, nonché gli enti privati *non profit* costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche,

compiti di formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari, per lo sviluppo di iniziative di informazione, sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze, e per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nonché con funzioni di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari, di promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze e di formulazione di proposte per favorire la messa in rete e l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati. è composto da rappresentanti di vari Ministeri, quali il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, quelli della salute, dell'ambiente del territorio e del mare, dello sviluppo economico e manca però il Ministero dell'istruzione. Voglio sperare che, considerate le implicazioni educative del provvedimento, si aggiunga un posto a tavola anche per una rappresentanza del MIUR

Le parti più complesse sono quelle che ci inducono anche ad ammettere una serie di ordini del giorno importanti, rinviando alla scrittura del scrittura del decreto legislativo la parte relativa al riuso dei prodotti farmaceutici. È stato svolto un buon lavoro, veloce, e credo che anche se il testo che uscirà da questa Camera non dovesse subire cambiamenti, il lavoro che abbiamo svolto è importante perché porta all'approvazione del provvedimento in tempi rapidi, che sono quelli che si aspettano

per il lavoro svolto e per le riflessioni che sono state avanzate su questo importante provvedimento che, a mio avviso, com'è stato giustamente detto, è una delle più belle e più concrete eredità del nostro Paese dopo l'Esposizione universale di Milano 2015. Abbiamo molto lavorato nei sei mesi di Expo e anche nei mesi successivi per finalizzare, il passo che compiamo definitivamente oggi con questa legge. Si tratta della traduzione operativa di principi fondamentali che abbiamo richiamato nel nostro lavoro, nella Carta di Milano, nel campo di relazioni internazionali che abbiamo sviluppato grazie all'Esposizione universale su una frontiera fondamentale come quella della lotta agli sprechi. Sarà sempre di più una delle grandi questioni internazionali di sostenibilità e competitività dei modelli di sviluppo e vedrà in particolare l'Europa e l'Italia, nel cuore del Mediterraneo, segnare sperimentalmente, con questa legge, alcune vie nuove di cittadinanza e di promozione delle buone pratiche. Questo è un grande tema che ci riguarda tutti. Ha un valore, com'è stato giustamente ricordato da tanti in quest'Aula, anche economico-finanziario tutt'altro che irrilevante, parliamo di più di 10 miliardi di euro di spreco alimentare nel nostro Paese, una cifra inaccettabile. Le norme che consolidiamo con questa legge ci consentiranno, a mio parere, di raggiungere l'obiettivo del recupero di un milione di tonnellate di cibo e di convertire questo spreco in donazione, così come abbiamo dimostrato di saper fare in questi anni, praticando la via della partecipazione consapevole a queste scelte, in particolare investendo sul sistema del terzo settore, sulle reti associative e sul protagonismo diffuso di responsabilità e cittadinanza di tanti.

raccontare anche fuori confine e che segna un discrimine profondo tra il modello italiano di lotta allo spreco alimentare e altri modelli. Noi qui misuriamo uno scarto e una differenza tra la via italiana alla lotta allo spreco alimentare e quella che hanno preso altri Paesi. Quello che confermiamo con questa legge è un modello promozionale, partecipativo, premiale e non punitivo; investe sulla cittadinanza responsabile, sulla consapevolezza diffusa, tanto delle aziende, quanto dei cittadini e delle famiglie e penso che dobbiamo tutti essere orgogliosi di aver contributo ad affermare questi elementi di novità. Credo che con questa legge potremo consolidare quel laboratorio che si è sviluppato, in particolare, in questi ultimi anni, con la grande consapevolezza che, per combattere lo spreco alimentare e lavorare sempre più e meglio sul versante del sostegno agli indigenti, servono tutti questi strumenti. Dobbiamo mettere in campo, come stiamo facendo, una pluralità di iniziative credo che la legge di oggi sia un fatto nuovo, molto importante per tutti noi. Toccherà a ciascuno esserne all'altezza anche nei prossimi mesi e quindi sviluppare più più avanti, oltre l'approvazione di questa legge, un campo di responsabilità e di impegni che sia all'altezza della discussione che abbiamo sviluppato e promosso con Expo Milano 2015. Questa è un'eredità concreta

1. Lo dico per cortesia nei confronti di quest'Assemblea: mi sarei aspettato che il Ministro restasse almeno per l'esame dei

Il nostro voto favorevole è motivato da una ragione molto semplice. Come già abbiamo argomentato precedentemente, chiediamo che tutto ciò che riguarda la materia farmaceutica sia espunto dal provvedimento, diventando oggetto di uno specifico

gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 8.0.1, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, per estraneità

di un tavolo con la GDO e le organizzazioni solidaristiche.

attraverso l'emendamento 3.203 si vuole introdurre, nei confronti degli operatori del settore alimentare, un vero e proprio obbligo, al posto della mera facoltà di cessione gratuita delle eccedenze alimentari. Questo allo scopo di rendere degne di un qualche rilievo le ricadute positive del provvedimento all'interno del territorio nazionale.

non si contempla la possibilità della cessione a titolo gratuito delle eccedenze che hanno un utilizzo a fini specialistici, per pazienti in in nutrizione domiciliare artificiale. Questi prodotti, che hanno un costo importante e un'utilità indubbia, vengono gettati e non hanno più la possibilità di essere utilizzati.

una semplice precisazione, che però è essenziale dal nostro punto di vista, ovvero che i prodotti trasformati debbono essere ceduti ai consumatori e agli utilizzatori finali in forma gratuita. Sembra una cosa da poco, ma siamo in un Paese che purtroppo ci ha abituato, anche nelle migliori circostanze, a fenomeni di degenerazione. Definiamo una specifica che, in maniera chiara ed evidente, determini la gratuità della cessione dei prodotti, affinché sia evitata in qualsiasi forma l'eventuale cessione a titolo oneroso o, addirittura, la reimmissione sul mercato del prodotto lavorato, quale potrebbe essere un pane trasformato che viene a diventare un prodotto differente ed è rimesso sul mercato. No, questo non può essere. Questa filiera deve definire in maniera

Signor Presidente, al fine di evitare potenziali deformazioni della *ratio* alla base del disegno di legge in esame, nell'emendamento 4.200 si ritiene opportuno specificare che anche i prodotti trasformati, ai sensi di quanto prescritto dell'articolo 4, devono essere ceduti in forma gratuita sempre in un contesto di solidarietà sociale.

la preminenza dell'attività del Ministero delle politiche agricole non possano che essere riconosciute in questo ambito, in questo campo e in questa funzione.

lo ritiri perché la forma più attenuata è quella che lui propone nell'ordine del giorno G9.200, del quale propongo una riformulazione.

obiettivi, impegna il Governo: a promuovere iniziative, in raccordo con il MIUR, volte a rafforzare il ruolo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella predisposizione di percorsi mirati, anche attraverso le istituzioni scolastiche, di educazione alimentare contro lo spreco». Sull'ordine del giorno G9.201 della senatrice Moronese il parere

«impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la pubblicizzazione delle informazioni utili, linee guida, iniziative istituzionali e di campagne informative in attuazione della presente legge, anche mediante una sezione *web* dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari».

Presidente, io sono abbastanza stupito, non voglio eccedere dicendo sconcertato o altro. Signor Ministro, il provvedimento è stato incardinato in Commissione agricoltura,

Presidente, alla luce di quello che ho appena detto, la ringrazio per avere sollecitato la mia risposta ma ovviamente questa non può che essere contraria. volevo solo tranquillizzare il senatore Candiani rispetto alla sua osservazione. Io credo che la proposta di riformulazione abbia un senso anche nelle dimensioni

Presidente, se si crede nel provvedimento, bisogna anche finanziarlo. Il provvedimento sta in piedi con un milione di euro. Sfido voi a ritenere che questa non sia una cifra simbolica.

nei confronti del Ministero e del Presidente del Consiglio dei ministri. Forse è l'ennesima occasione per fare un *tweet* pre-estivo del tipo: «Abbiamo approvato la legge sugli sprechi alimentari».

anche del mondo economico, che deve tener conto poi di ciò che stiamo approvando. È facile dire che si fanno le leggi se poi sul territorio qualcun altro paga i conti. Signor Presidente, volevo rassicurare il senatore Candiani che tutte le attività nelle scuole vengono sempre e comunque fatte a costo zero. Questa è la caratteristica. Anche questa sarà

quindi con uno spirito di fondo che dovrebbe essere quantomeno riconosciuto e apprezzato dal Governo, non tenga conto anche della liceità da parte di questa Camera di apportare delle modifiche

Lettieri)*. Noi stiamo approvando un provvedimento nel quale crediamo: l'abbiamo detto prima nella discussione generale

su questo articolo alla Camera sono stati approvati dei nostri emendamenti che almeno hanno consentito di fare in modo, per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci, dei farmaci, che le associazioni che ne avranno disponibilità accompagnino l'uso dei farmaci con le debite professionalità. Non si usano i farmaci se non si ha la professionalità e la capacità di distinguere: non è un pezzo di pane secco che si può dare a una persona o un'altra. Almeno quella misura Ma insistere ancora con questo atteggiamento che cosa vi produrrà alla fine? Avrete approvato il provvedimento? Va bene, ma qual è lo spirito con cui lo avrete approvato? È quello di voler fare l'ennesima dimostrazione che avete i numeri per farlo? Francamente non è il caso e si perde anche un'opportunità per dare un segno distintivo di cosa sa fare la politica oltre gli schieramenti.

la sensazione al Paese che il provvedimento viene approvato e consegnato per rappresentare la risposta ad un bisogno. Sarebbe tutto vero e tutto giusto se non ci fosse una semplice osservazione, ossia il fatto che paradossalmente un disegno di legge, uno dei pochissimi di iniziativa parlamentare, viene strozzato

Io personalmente anticipo quello che poi in modo più dettagliato esprimerò in dichiarazione di voto: questa è la mortificazione della democrazia parlamentare. Seconda considerazione per quanto riguarda l'articolo 15 (così assorbo dentro questo intervento le mie considerazioni). Si perde un'opportunità, e lo ha ricordato molto giustamente, pacatamente e propositivamente il collega Candiani da ultimo con il suo intervento: l'atteggiamento delle opposizioni è finalizzato a portare un segno di miglioramento al testo del provvedimento, ma la risposta è assolutamente incoerente ed irresponsabile.

senza rendersi conto di cosa si sta votando; poi, *ex post*, si deve dare conto al Paese di provvedimenti assolutamente inadeguati. Si dice che il meglio è nemico del bene. Qui sorride la mia amica e collega Emilia De Biasi, con la quale abbiamo un dibattito politico vivace in 12a Commissione, ma poi - vivaddio - c'è una convergenza, perché c'è il senso di una maturità politica che ci porta a convergere su tanti provvedimenti. con qualche imbarazzo colleghe e colleghi del Partito Democratico in Commissione sanità che lanciano la pietra e nascondono la mano, e poi alla chetichella scompaiono tutte quelle granitiche affermazioni che si sciolgono come neve al sole perché la disciplina di partito dice che bisogna approvare il provvedimento così come è giunto dalla Camera. Ma questa non è democrazia parlamentare, caro Presidente. L'articolo 15 per competenza di materia è stato sottoposto alla valutazione della 12a Commissione. Nel parere espresso dalla 12a Commissione,

rilevato che il testo dell'articolo 15 summenzionato appare connotato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune, tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alle disposizioni e da far supporre senza precisare che vi è la necessità che la predetta attività debba essere svolta a cura di personale abilitato alla professione di farmacista (...)» - altro elemento nella narrativa del provvedimento - e si conclude poi con il parere favorevole. Ma qui c'è un parere

che recupera il testo del disegno di legge a mia firma, che la collega della Camera ha pensato di asportare dalla competenza del Senato, che lo aveva già incardinato, lo aveva già votato e sull'argomento aveva anche audito il direttore generale dell'AIFA, con tutte le osservazioni e i suggerimenti correttivi che avevano formato oggetto di emendamenti.

sciatto, disordinato e anche arrogante di legiferare. Questo è il motivo per il quale chiedo la soppressione dell'articolo 15 e, in via subordinata, chiedo l'approvazione dei correlati emendamenti che ne modificano il contenuto,

e una donazione che non dà nessuna possibilità di essere garantita da un professionista della salute, nell'atto e nel momento in cui c'è bisogno di questo aiuto. aiuto. Sostanzialmente prevediamo che non ci sia davvero una figura professionale qualificata, che possa aiutare chi ha bisogno a sapere se un tale farmaco è davvero necessario a quella persona

con gli emendamenti in esame vogliamo solamente cercare di fare del diritto alla salute una cosa vera e non un momento fasullo. Penso, in generale, che, quando abbiamo bisogno di un aiuto, sia sempre necessaria una persona qualificata, e a maggior ragione, se l'aiuto serve per una scelta che influisce sulla nostra salute, abbiamo bisogno di avere la certezza

ma perché tutti i cittadini davanti alla salute - come dice la Costituzione - devono essere uguali e, quindi, i diritti di chi paga devono essere gli stessi di chi riceve un farmaco. Nell'illustrazione spero davvero che possano essere recepiti i nostri emendamenti e che chi ha bisogno possa essere trattato come chi paga un servizio nel Servizio sanitario nazionale.

Senatore Volpi, lasci concludere

Signor Presidente, io sono sempre estremamente gentile e cortese ed entro sempre in punta di forchetta. Questo è un tema estremamente delicato e vorrei terminare il mio ragionamento.

un farmaco è il medico e chi distribuisce il farmaco è normalmente, anzi per legge, il farmacista.

chi prescrive il farmaco - quindi anche in questo caso - è il medico e chi lo distribuisce deve essere sempre un farmacista. Infatti, nel disegno di legge che noi avevamo incardinato - e che era alla fine del suo percorso legislativo,

le associazioni, le ONLUS, avrebbero collaborato con le associazioni territoriali dei farmacisti affinché fosse sempre un farmacista a distribuire il farmaco.

abbia consapevolezza di ciò che ha affermato. Ella ha asserito Ella ha asserito che il Governo, nell'emanare il decreto attuativo sull'articolo 15 in discussione, avrebbe dato ampie garanzie sul fatto che avrebbe precisato le figure addette alla distribuzione dei farmaci e quant'altro. pare, però, che, quando si conferisce una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni di legge, vi siano delle regole che non possono essere superate. La delega deve indicare esattamente i limiti

quello che deve scrivere nel decreto attuativo. Per carità, tutta la fiducia al Governo la esprimiamo anche quando diamo il nostro voto di fiducia, ma attenzione: in questo caso stiamo parlando di qualcosa di estremamente delicato. delicato. Si parla di figure che devono distribuire farmaci «ove necessario», e quindi si danno i più ampi spazi per fare di questo provvedimento qualcosa che potrà essere gestito a uso e consumo non so di chi.

fare più attenzione nel prestare garanzie fiduciarie a un Governo che non intende correggere il testo o precisarlo nella sede naturale, e cioè in quest'Aula, ma che pensa di riservarsi

il decreto sarà efficace del nostro Paese e il danno sarà divenuto irrecuperabile. Questa è la sede in cui ancora si può recuperare. Invito allora a riflettere su tale punto e a consentire a quest'Assemblea l'esame del provvedimento, apportando quelle correzioni, in particolar modo all'articolo 15,

Signor Presidente, rubo solo qualche minuto. È chiaro che, quando un provvedimento arriva in Assemblea, non tutti l'hanno istruito - succede anche a noi per i provvedimenti delle altre Commissioni - e quindi è normale che

Ci siamo trovati, signor Presidente, di fronte a una situazione molto sgradevole, perché si è messa in discussione la leale collaborazione tra i due

assolutamente vero, tant'è vero che abbiamo scelto tant'è vero che abbiamo scelto deliberatamente di inserire questa valutazione nel parere: elemento di solito non rituale, ma a noi è parso che ci fosse un legame forte da evidenziare proprio su questo punto.

e mi prendo la responsabilità di quello che dico - o se demandare non necessariamente a un'indicazione al Governo, ma a un disegno a un disegno di legge in grado di completare le lacune presenti - un disegno di legge ripreso esattamente dal relatore, senatore D'Ambrosio Lettieri, dalla senatrice Bianconi e dalla sottoscritta

secondo quanto scritto nell'articolo 15, riservandoci però una parte di approfondimento nel disegno di legge che rimane comunque in vigore.

nell'esame del disegno di legge che è già incardinato e che prevede di mettere a posto le cose sicuramente meglio di quanto abbia fatto la Camera dei deputati. *(Applausi

con questo emendamento chiedevamo una cosa proprio banale, che dimostra la volontà di non venire incontro alle opposizioni. Chiedevamo che presso il Ministero della salute fosse attivato un sito nel quale poter far affluire le donazioni su una specie bacheca e, quindi, mettere in contatto chi donava con chi eventualmente su quel sito del Ministero della salute poteva trovare

so che il Ministero disciplina in un sito *ad hoc* la mia donazione ma, soprattutto, quello che mi interessa è che chi cerca qualcosa sa dove andare a cercarlo.

quando c'è la donazione di un farmaco, sia garantita quella catena di sicurezza, prevista dal sistema sanitario italiano, che possa dare la possibilità anche a chi non ha i soldi ma ha bisogno di un farmaco di avere le stesse garanzie di chi paga.

Mi riferisco soprattutto, prendendo in prestito l'emendamento del senatore Mandelli, alla questione del personale sanitario, che è una figura ben definita dalla legge e non è solamente

il fatto che dire che le società assistenziali sono equiparate al consumatore finale significa che il consumatore finale è il cittadino che mette il farmaco nel proprio armadietto

siamo d'accordo; ma dove non è necessaria, il farmaco viene distribuito a pioggia, creando un grande problema di sicurezza che la stessa Presidente ci ha detto che bisogna sistemare il più presto possibile. Noi ci auguriamo che il

che non sia l'infermiere o altro, qualunque infermiere potrà fare ricorso avverso quel decreto e non ci sarà tribunale amministrativo che non gli darà ragione. L'eventuale decreto attuativo che vorrà specificare che la distribuzione debba essere fatta da medici o da farmacisti, e non già anche da altre figure professionali, contrasterà con il contenuto della delega. Io ritengo sin d'ora di poter affermare serenamente che qualsiasi tribunale amministrativo italiano accoglierà il ricorso, perché riterrà che il decreto attuativo ha limitato ciò che, invece, la legge delega aveva ampliato. Per queste ragioni solleciterei l'approvazione dell'emendamento 15.11 e non già eventuale trasformazione in ordine del giorno, come ha suggerito anche il capogruppo Barani.

Presidente, mi rendo conto che la curva di attenzione declina il brusio prevale sulla necessità di approfondire alcuni passaggi esposti in punta di diritto dal collega Falanga.

consegnare la responsabilità a rimettere le carte in regola al decreto del Ministro pone la domanda del perché non possiamo fare oggi

l'utilizzazione e i requisiti. Mancano i riferimenti alla modalità di cessione all'utilizzatore finale e non si potrà fare,

consenta di evitare il ripetersi di questo teatrino che è grave e avvilente non solo per noi, ma per la democrazia del nostro Paese.

abbassate il tono di voce, così posso sentire la relatrice. BERTUZZI, *relatrice*. Accreditato alla distribuzione dei farmaci. Il titolo per l'accredito alla distribuzione è anche abilitato alla professione di farmacista, io consiglierei un'espressione che è anche presente nei testi, ossia: «la distribuzione secondo la normativa vigente»,

Il parere della 12a Commissione è puntuale nei termini, esaustivo nei contenuti e risolutivo della questione che stiamo valutando. oltre a essere un parere reso alla 9a Commissione, diventa anche un atto di impegno del Governo ad adeguarsi alle indicazioni della Commissione, che per competenza ha espresso il parere, credo che

la riformulazione è quella che abbiamo realizzato con il contributo della relatrice e della Presidente della 12a Commissione. Oggi non c'è la possibilità che nasca *ex novo* un ordine del giorno che riproduca il parere da lei citato. Se lei accetta la riformulazione,

Il Gruppo Forza Italia non può che essere contrario all'approvazione di questo articolo, perché è la dimostrazione del fatto che pur quando un provvedimento non ha nessuna connotazione ideologica,

che lo si guardi da una parte o dall'altra di uno schieramento. Occorre solamente cercare di aiutare i tanti italiani che rinunciano ad una cura perché non se lo possono permettere. Questo era il senso con cui abbiamo affrontato l'articolo 15 e il senso che avremmo voluto vedere nel lavoro della Commissione. Invece, siccome bisogna fare presto, non c'è spazio e non c'è tempo per fare diversamente, andiamo a fare un bel

che, ricordo a me stesso, recita: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo; considerato che il disegno di legge persegue la condivisibile finalità di limitare gli sprechi e incentivare la donazione e la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale; rilevato che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di inserire nel testo disposizioni "in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali" (così recita la rubrica dell'articolo 15), malgrado in proposito presso il Senato fossero in corso d'esame, dal 2 marzo 2014, disegni di legge specifici, giunti alla fase emendativa (disegni di legge n. 1092 e connesso)»; perché resti agli atti: «rilevato che il testo dell'articolo 15 summenzionato appare connotato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alle disposizioni e da far supporre un non adeguato livello di approfondimento istruttorio». rilevato che, per ciò che attiene alla cruciale attività di dispensazione dei farmaci oggetto di riutilizzo, il testo pone la condizione, alquanto generica che le Onlus dispongano di "personale sanitario", senza precisare che vi è la necessità che la predetta attività debba essere svolta a cura di personale abilitato alla professione di farmacista». Presidente, questo è il parere redatto dalla 12a Commissione e, a fronte di questo parere, sono stati proposti emendamenti che la maggioranza oggi qui, in Aula, ha respinto. Io mi chiedo, vi chiedo, con quali responsabilità licenziate questo testo di legge. Abbiamo proposto una cosa molto semplice: si faccia una ottima legge sullo spreco alimentare, ma non si mescolino i farmaci con gli alimenti, perché chi si nutre di farmaci va al creatore.

Signor Presidente, in dissenso dal voto dichiarato dal senatore Mandelli, cosa che naturalmente mi costa non poco, dichiaro che non parteciperò al voto su questo articolo, per un motivo molto semplice. In questa XVII legislatura, che passerà alla storia per il massacro della Costituzione, o sotto forma di riforma o sotto forma di interventi anomali da parte del Parlamento, mi era capitato di ascoltare di tutto in ordine al bicameralismo. Ma questo mi era sfuggito: bicameralismo imperfetto a tappe.

questa fretta di legiferare così male, non tenendo conto della normativa già esistente e non armonizzando la norma

Siamo talmente abituati ai decreti d'urgenza *mix,* che evidentemente non ci rendiamo più conto di cosa sia razionale e

voi abbiate letto bene l'articolo 16 e soprattutto se lo abbiano letto coloro che in quest'Aula svolgono le funzioni di vestali della legalità e di affermatori del sospetto. Avete letto che sono esonerate dalla comunicazione alla Guardia di finanza le

che si apprestano a contabilizzare 14.500 euro per ogni spedizione e che fanno 10, 15, 20 spedizioni mettendo in piedi *business* particolari soprattutto sui prodotti farmaceutici. non si può stabilire un limite al di sotto o al di sopra del quale si devono fare tali comunicazioni. Queste comunicazioni devono essere fatte per ogni partita di merce che va a cedersi gratuitamente. Il limite dei 5.000 euro mi viene ispirato da quello che tutti noi abbiamo nel dichiarare i contributi per quanto riguarda gli aspetti della campagna elettorale.

con la compiacente prestazione d'opera di banchi alimentari non proprio perfettamente in linea con la nobile filosofia di questo provvedimento, io davvero mi domando come possiamo accettare

minimamente degnati di rilevare che questa è una voragine che si apre nelle possibili truffe al commercio e anche all'evasione fiscale. È una voragine che si apre.

opportune modifiche in maniera tale che questa attività non si presti al benché minimo aspetto di truffa o di elusione fiscale o a qualsiasi tipo di malversazione, cosa che invece accadrà sicuramente. Veramente non capisco come possiate stabilire un limite di 15.000 euro all'obbligo di comunicazione sul trasferimento a cessione gratuita di questi beni; è veramente incredibile che non vi siate accorti di questa cosa. Pertanto voterò sicuramente contro l'articolo 16.

è stato esaustivo, puntuale e dettagliato nel descrivere i punti di forza di questo disegno di legge e nell'evidenziare la necessità che fossero un patrimonio legislativo che, ancorché tardivamente, giungesse a beneficio della nostra comunità. In particolare, ha puntualizzato come e quanto questo disegno di legge intercetti un bisogno diventato sempre più impellente, anche in coincidenza con la situazione gravissima della crisi economico-finanziaria che attanaglia da tanti anni il nostro Paese. Quindi, sostanzialmente, ha spiegato come e quanto il concetto della povertà alimentare non sia purtroppo limitato soltanto ad alcune parti del mondo, ma sia un fenomeno esteso, che riguarda oggi 53 milioni di di cittadini europei che fanno fatica a mangiare un pasto completo ogni giorno. In Italia, in cinque anni, sono più che raddoppiate le persone che non possono più permettersi una dieta equilibrata. Questa è una materia nella quale si registrano dei veri e propri paradossi. Un paradosso è che, nel 2011, noi abbiamo avuto una notizia che è, al tempo stesso, una bella e una brutta notizia. La bella notizia è che il numero delle persone che muoiono di fame si è ridotto; la brutta notizia è che sono aumentate le persone che muoiono per iperalimentazione, ovvero per le patologie che derivano dagli eccessi alimentari. Quindi siamo contenti che diminuiscano i denutriti, ma siamo preoccupati per il fatto che aumentino le persone in sovrappeso e gli obesi. Questo è il paradosso che si registra anche nel dibattito, nell'approfondimento, nelle ragioni che ruotano attorno a questo disegno di legge. Il problema degli sprechi alimentari infatti riguarda tutto il mondo. Secondo i dati della FAO, ben un terzo del cibo del mondo finisce sprecato; parliamo di oltre un miliardo e 300 tonnellate di spreco, che rappresentano sostanzialmente la quantità di cibo necessaria per sfamare un miliardo di di persone, che oggi soffrono la fame perché non hanno accesso sufficiente alle risorse alimentari. Solo nei Paesi industrializzati vengono buttate via oltre 220 milioni di tonnellate di cibo E ancora, ogni anno finiscono tra i rifiuti dai 10 ai 20 milioni di tonnellate di prodotti alimentari, per un valore stimato in oltre 30 miliardi. Quindi ci sono aspetti di natura etica, di natura culturale e anche problemi, soprattutto di natura sociale, dovendosi necessariamente rimettere in equilibrio quel forte sbilanciamento, che esiste e che diventa odioso per i livelli gravissimi di discriminazione, che sta nelle disuguaglianze Ma ci sono altri fattori che devono essere tenuti a mente e che il mio collega senatore Liuzzi ha ricordato. La riduzione degli sprechi alimentari coincide con un interesse dell'ambiente, perché diminuisce il volume dei rifiuti. E ancora, combattere lo spreco alimentare è importante anche perché contenere l'impatto sulla biodiversità della della produzione massiva di alimenti diventa un vero e proprio problema, una sorta di emergenza. dell'espansione agricola e delle coltivazioni estensive sulla frammentazione degli *habitat* e sulla perdita della biodiversità sono tali che appare veramente inconcepibile e inaccettabile che una parte rilevante di quanto prodotto venga poi gettato. Si potrebbero ancora ricordare altri punti che rappresentano elementi di forza per condividere questo provvedimento. Invece la nostra posizione, purtroppo, è di grande perplessità e anche di rammarico. nella democrazia parlamentare l'Aula svolge una funzione fondamentale. Nell'Aula si svolge il confronto tra le diverse posizioni, quando il confronto si affranca da speculazioni, da nodi ideologici che talvolta allontanano la politica dal bisogno della comunità e creano un corto circuito tra la piazza e il palazzo che determina situazioni assai gravi che avremmo potuto ben superare se solo ci fosse stato un atteggiamento diverso da parte della maggioranza e di questo Governo che la maggioranza sostiene. Cicerone, nel «De natura deorum», quando parla dei pitagorici che si rivolgono al loro maestro, ricorda che

così è stato stabilito e così si deve fare. Una situazione grave quella che si è verificata ieri con il 53° voto di fiducia oggi con un paradosso: uno dei pochissimi disegni di iniziativa parlamentare viene consegnato all'approvazione attraverso la strada stretta e tortuosa di un dibattito fine a se stesso, inutile e ozioso che ha aperto la porta, quando è andata bene, a qualche garbata e generosa concessione

finalità ostruzionistiche né erano finalizzati a stravolgere il senso del testo che ci è giunto dalla Camera. Gli emendamenti erano pochi e tutti orientati a sostenere con coerenza, con forza e con ragionevolezza un testo sul quale si è registrata, tutto sommato, una discreta condivisione. l'*ipse dixit* ha elevato il livello di arroganza, di prepotenza, di supponenza del Governo e della maggioranza e non si è potuto fare quello che sarebbe stato necessario fare. [**Presidenza

- del suddetto articolo - appare connotato da criticità relazionali, imprecisioni e lacune, tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alla disposizione e da far supporre un non adeguato livello di approfondimento istruttorio». E che si fa? Si delega al Governo il compito di porvi rimedio. Non si affida all'Assemblea, non si affida alla democrazia parlamentare, alla propositività dell'emendamento la correzione di un testo che è decretato come insufficiente, inadeguato e lacunoso, ma lo si vota con l'applauso, con il sorriso, con il compiacimento, con l'autocelebrazione, per dover correre domani in piazza a rappresentare una verità che non c'è, la verità che si porta un provvedimento che è risolutivo

che porta il Gruppo dei Conservatori e Riformisti a sottolineare l'assoluta irresponsabilità del Governo e della maggioranza e necessariamente a esprimere un voto di astensione che - torno forse sarebbe stato necessario, un voto contrario al contenuto della legge. È, invece, un voto attraverso il quale si intende esprimere la censura rispetto al metodo con cui, in quest'Aula, la la maggioranza e il Governo impongono la loro volontà e il loro *Diktat* ferendo la democrazia. Signor Presidente, voteremo questo provvedimento perché colma un vuoto normativo e va a incidere positivamente su una situazione a due facce. Da una parte, abbiamo un grande fenomeno in Italia, come in tutti gli altri Paesi dell'Occidente, di sprechi alimentari, vale a dire di prodotti che ai vari stadi della filiera vengono accantonati,

molto anche il comportamento delle stesse famiglie. Tutto ciò ha una ricaduta economica negativa sull'intero funzionamento della filiera. Dall'altra parte, c'è una fascia della popolazione, purtroppo sempre più ampia, che versa in condizioni di povertà assoluta. Le statistiche sono impietose: nella sola Unione europea si sprecano circa 90 milioni di tonnellate di cibo e il 55 degli sprechi di alimenti sarebbe ancora idoneo per il consumo umano. In Italia lo spreco alimentare ammonta a circa 6 milioni di tonnellate, il cibo sprecato è di 108 chilogrammi *pro capite* e ogni anno una famiglia media getta via 450 euro.

In un anno si potranno recuperare in Italia 1,2 milioni di tonnellate di derrate alimentari che rimangono ora sui campi, altri 2 milioni di tonnellate di cibo che provengono dall'industria agroalimentare e più di 300.000 tonnellate provenienti dalla Un terzo del cibo prodotto annualmente nel mondo viene gettato tra i rifiuti e corrisponde a quattro volte la quantità necessaria per nutrire gli affamati del Pianeta, che sono 868 milioni di persone. Se è facile produrre cibo, è invece molto più difficile conservarlo e trasferirlo, anche se le nuove tecnologie permettono sempre più di migliorare la conservazione dei prodotti. Da un punto di vista quantitativo, non c'è una grossa differenza tra lo spreco nei Paesi industrializzati rispetto a quelli in via di sviluppo, se non nell'ultimo passaggio, che è quello dello spreco domestico. Nei Paesi in via di sviluppo la difficoltà di conservare il cibo implica una riduzione ai minimi termini della produzione di spreco, mentre nei Paesi industrializzati, per una questione di stile di vita, lo spreco domestico è altissimo, pari al 42 per cento dello spreco totale. Bisogna, quindi, da un lato, offrire ai Paesi in via di sviluppo soluzioni a livello tecnico per una migliore conservazione del cibo - ed è proprio ciò che la FAO ha deciso di fare negli ultimi anni investendo sul confezionamento - mentre, dall'altro, è necessario agire nei Paesi industrializzati sull'educazione e sull'informazione dei cittadini, che non a caso sono parti integranti di questo provvedimento. Una visione d'insieme della filiera consente di individuare in maniera incisiva i passaggi più critici in termini di perdite e d'impatto ambientale. In Italia alcune grandi imprese hanno aderito a un progetto per calcolare l'impatto ambientale del proprio prodotto lungo tutta la filiera. È il momento della produzione degli ingredienti, all'inizio quindi della filiera, quello che pesa di più sull'ambiente, mentre la distribuzione, passaggio finale, vi incide in maniera minima. Non è, quindi, solo un problema di distribuzione. Per non sprecare è importante essere consapevoli dell'impatto sull'ambiente di ciascun prodotto, così come è fondamentale la prevenzione nella produzione degli sprechi. Per quanto riguarda il recupero delle eccedenze e della loro cessione, in Italia da un punto di vista fiscale, con il decreto legislativo n. 460 del 1997 e con la legge n. 444 del 2007, sono previste delle agevolazioni per chi cede gratuitamente le eccedenze a favore delle ONLUS. Restano però alcuni limiti facilmente superabili che possono rendere meno complessa la procedura. Anche in questa direzione, il provvedimento che stiamo per approvare compie un indubbio passo in avanti. Sulla normativa ambientale è giusto intervenire con la politica di incentivi per rafforzare le azioni di recupero e di riutilizzo e ridurre quanto più possibile la produzione di rifiuti. Molti Comuni lo hanno già fatto, prevedendo - ad esempio - uno sconto sulla tassa dei rifiuti per le aziende impegnate nel recupero e nel riciclo. Di grande importanza è anche l'aspetto igienico-sanitario, perché è molto difficile recuperare e riutilizzare l'invenduto. necessario intervenire per armonizzare la normativa igienico-sanitaria attraverso linee guida chiare e specifiche per le organizzazioni *non profit* impegnate nel recupero delle eccedenze alimentari. Dunque, la semplificazione e l'armonizzazione di norme e procedure a livello nazionale permetteranno un maggiore ricorso alle pratiche virtuose di recupero. Mi avvio a concludere. Il provvedimento in esame dà una sistemazione normativa organica a tutti gli aspetti Vengono semplificate le procedure di donazione e distribuzione agli indigenti delle eccedenze alimentari. Chi donerà avrà incentivazioni fiscali e potrà ottenere uno sconto sulla tassa dei rifiuti proporzionale alla quantità di cibo donato. Si tratta di una da tempo invocata dagli operatori del settore. Viene estesa la platea delle associazioni *non profit* coinvolte e sono istituiti diversi fondi per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti per incentivare la riduzione dei rifiuti. Noi crediamo, a questo proposito, che puntare sugli incentivi sia stata una strada più convincente di quella percorsa in Francia, che impone unicamente regole e sanzioni alla grande distribuzione, non tenendo conto che le principali fonti di spreco alimentare sono i nuclei familiari. Quindi l'obiettivo, anche in futuro, dovrà essere mettere sempre più in sintonia, da un lato, l'attività delle organizzazioni caritative e, dall'altro, la disponibilità degli sprechi alimentari, soprattutto quelli che si determinano nello stadio della distribuzione. Per questi motivi, il Gruppo Alleanza

Signor Presidente, ci saremmo aspettati una maggiore attenzione e apertura da parte della maggioranza nella valutazione degli emendamenti al provvedimento

Che l'avessimo ben chiaro e, soprattutto, che avessimo intenzione di sostenerlo è stato chiaro dall'approvazione degli articoli, nonostante la bocciatura degli emendamenti di buon senso proposti.

«rilevato che il testo dell'articolo 15 summenzionato appare connotato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alle disposizioni e da far supporre un non adeguato livello di approfondimento istruttorio». Mescolare il tema dei farmaci con la necessaria attenzione a non sprecare gli alimenti significa veramente mescolare le mele con le pere, utilizzando un vecchio detto. Lo dico a qualche senatore che precedentemente aveva l'ambizione di rappresentare gli orientamenti di voto della Lega Nord. Noi siamo responsabili e consapevoli la maggioranza forza la mano per portare a un voto, indipendentemente e indifferentemente dal nostro consenso o dissenso.

portando in detrazione l'IVA o andando a recuperare costi che altrimenti andrebbero dispersi assieme alle derrate alimentari che invece vengono destinate ancora alla filiera alimentare e non alla discarica.

di inserire il recupero dei farmaci e la distribuzione degli stessi in una maniera che non esito a definire superficiale all'interno di questo provvedimento.

porterà le associazioni che recupereranno i farmaci per la distribuzione gratuita a doversi avvalere di personale sanitario. Non è sufficiente,

Questo nonostante la retorica del ministro Martina e del Presidente del Consiglio dei ministri ci abbia abituato, nei mesi passati, a sentirci raccontare che da Expo sarebbe nata una nuova pagina per l'agroalimentare italiano e, anche in questo caso, per la battaglia nei confronti dello spreco di cibo. A quanto pare, avete fatto passerella tagliando i nastri, dimenticando che questo obiettivo deve essere attuato,

e quello che invece è dovuto a modalità di mercato che normalmente vengono definite consumistiche. Occorre crescere, occorre investire perché ci sia un aumento di consapevolezza da parte dei cittadini a tutti i livelli. proposito, purtroppo, non ci soddisfa la misera dotazione prevista da questo provvedimento: inserire in un provvedimento così importante un milione di euro per sviluppare la politica del risparmio, della conservazione degli alimenti e per combattere gli sprechi alimentari su tutto il territorio nazionale in un anno, appare veramente cosa risibile. Questo dà un'idea della necessità, da parte del Governo, di chiudere l'approvazione del provvedimento, di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri la soddisfazione del solito *tweet*, rinviando invece la concretezza e la solidità del provvedimento che, privo di finanziamenti, avrà ovviamente Per questi aspetti non siamo soddisfatti, ma siamo consapevoli che il provvedimento debba essere approvato, perché, nonostante tutto,

vi avesse indicato le criticità e nonostante gli emendamenti presentati in Assemblea avessero individuato delle vie di uscita alternative. Sosteniamo la parte relativa alla necessaria politica contro gli sprechi alimentari e lasciamo a voi l'onere di avere sottovalutato gli aspetti relativi alla diffusione, temo poco controllata, dei farmaci recuperati e rimessi in distribuzione a chi non ha a disposizione un farmacista o un medico a cui potersi affidare.

ha espresso bene anche il senso del provvedimento e mi limito a rimarcare alcuni concetti generali, che ritengo importanti e in particolare il fatto che faccia seguito all'Expo di Milano e alla Carta di Milano, che io stesso, come molti altri colleghi,

quasi per caso e oggi molto strutturata, che raccoglie 2.000 tonnellate di alimenti all'anno, che altrimenti finirebbero nei cassonetti, e assiste ogni giorno centinaia di famiglie bisognose. Quindi, si tratta, di fatto, di una prassi che esiste già ed è bene averla in qualche maniera regolamentata e istituzionalizzata. la prima parola d'ordine che il disegno di legge deve avere è quella della semplicità e della accessibilità. Non si tratta di una legge nata per creare nuova burocrazia o sovrastrutture, né mi auguro per creare nuovi uffici, ma per rendere possibile una pratica che dovrebbe essere propria di ogni

comunque è buona, pur di raggiungere l'obiettivo, che oggi è duplice. Siamo di fronte a dati preoccupanti, diffusi dalla FAO, dalla Commissione europea e da alcuni istituti di ricerca, che ci dicono che oggi aumentano gli sprechi alimentari ma aumenta anche la povertà. Quindi, di fatto è una contraddizione che abbiamo il dovere morale, oltre che civile, di sanare. Quindi, oggi la lotta contro ogni tipo di spreco deve essere un obiettivo fondamentale l'educazione civica per un uso consapevole delle risorse altrettanto. Spetta a questo Parlamento cercare di dare un aspetto un aspetto normativo che renda più facile quanto dovrebbe avvenire nel comportamento di ogni giorno. All'interno di questo provvedimento vi sono molti aspetti positivi: da quelli educativi

Mi piace anche la semplificazione normativa per i produttori e distributori, che cerca di rendere ufficiale il concetto di gratuità e che va contro ogni tipo di speculazione. Altrettanto positivi trovo gli incentivi fiscali, che vanno dalla detraibilità e deducibilità di alcuni oneri per i distributori, come la possibile riduzione delle tariffe sui rifiuti per chi porta avanti queste pratiche. Certamente, la la sfida molto più importante, che va oltre questa legge, è quella che ci impone di rivedere gli stili di vita e di riconsiderare i modelli di consumo. La sfida è favorire la chiusura delle filiere, così che queste siano ad alta recuperabilità.

la protezione ambientale e il fatto che, comunque, produrre rifiuti e non recuperarli porta ad aumentare il costo della raccolta dei rifiuti e i relativi problemi di inquinamento. Altrettanto condivisibile è il fatto che quando gli alimenti non possono essere utilizzati per alimentazione umana siano recuperati per alimentazione animale o comunque per recupero energetico o, in ogni caso, per il riciclo. riciclo. Devono poi essere coinvolti in queste politiche oltre alle scuole tutti gli enti locali. Il mondo del volontariato è assolutamente indispensabile.

evitare il dramma che la burocrazia renda inefficace un provvedimento che, invece, vuole mettere in campo procedure efficienti e accessibili a tutti. Sicuramente vanno coinvolti gli operatori. operatori. Concludendo, questo non è un provvedimento facile, né di facile applicazione, ma comunque dovrebbe divenire una prassi costante. Mi auguro che il Governo riesca a renderlo concreto attraverso decreti semplici da applicare.

discusso è un provvedimento che parla dei limiti e delle contraddizioni della nostra società, del nostro modo di produrre e di consumare; è un disegno di legge che parla anche alle generazioni più giovani, molto attente alla salvaguardia del pianeta e quindi all'impatto ambientale di ogni nostra scelta, agli sprechi di risorse, alla coerenza parte da finalità condivisibili, ma tutto il testo vola molto alto e demanda di fatto ogni applicazione pratica al tavolo di coordinamento previsto all'articolo 8, che rischia di diventare un grande contenitore che produrrà qualche proposta ipermediata con tempi assai lenti, ma i ritardi accumulati in questi anni in realtà richiedono di intervenire in maniera rapida e determinata. L'intero testo è per noi un compromesso al ribasso rispetto a quanto già da anni avviene all'estero e che gli stessi disegni di legge racchiusi in questo unico testo in realtà hanno rappresentato. Il testo si pone l'obiettivo pratico di rendere possibile quanto oggi è di fatto vietato, ovvero regalare cibo e medicinali scaduti al fine di riutilizzarli e non farli andare perduti, ma è molto distante da quello che servirebbe in concreto: non prevede obblighi specifici, come ha invece scelto di fare la Francia, per la grande distribuzione

che devono destinare le eccedenze ricevute in forma gratuita e principalmente a persone indigenti. Se crediamo davvero nell'importanza di combattere lo spreco, servono obblighi definiti per tutti gli operatori, da quelli delle grande distribuzione a quelli al dettaglio, come avviene in molti altri Paesi europei, a partire dalla Danimarca, dove è fatto obbligo a tutti gli operatori - anche al dettaglio - del settore alimentare e a tutte le ristorazioni di conferire, al termine della giornata di lavoro, tutti gli avanzi in appositi sacchetti stagni, a prova di acqua e di altri agenti, fuori dai negozi.

che non può funzionare se non si fa educazione alimentare ed educazione al consumo consapevole. Tutto questo può funzionare solo se si coinvolgono gli studenti e gli insegnanti, quindi se si cambia il modello di sviluppo e di consumo. importante fare in modo, sulla base degli ordini del giorno approvati, che le Regioni possano stipulare accordi con i soggetti delle grande distribuzione per lo sconto sui prodotti in scadenza, che è estremamente diffuso in Europa (penso alla Francia, alla Svizzera, alla Germania, al Regno Unito) e che è il passaggio meno costoso e più immediato per favorire l'utilizzo del cibo prima della scadenza. Sarebbe stato opportuno prevedere il recupero di risorse importanti per garantire la promozione e l'attuazione di questo disegno di legge, come la tassazione delle bibite che contengono elevati livelli di zucchero, dannosi per gli adulti L'approvazione di un ordine del giorno sull'utilizzo di un'*app* per la circolarità della distribuzione delle eccedenze apre ovviamente ad enormi potenzialità, che permettono anche ai cittadini di mettere a disposizione il cibo in scadenza con una distribuzione a rete, proprio come avviene in Danimarca. Regalare, come avviene in moltissimi casi virtuosi, pane, pizza o paste a fine giornata da parte dei panifici o delle pasticcerie a singoli o organizzazioni sulla base di conoscenze o relazioni che le organizzazioni hanno instaurato da anni è una pratica che, proprio con la sperimentazione di una *app* gestita dal pubblico,

Per noi di Sinistra italiana il ruolo del pubblico dovrebbe essere quello di favorire questo scambio e premiare i cittadini in vari modi, ad esempio con lo sconto sulla tassa dei rifiuti per chi partecipa in maniera costante ad iniziative di riutilizzo e di messa in rete del cibo in scadenza. È invece prevista nella legge solo la riduzione sulla tassa dei rifiuti per le attività non domestiche relative ad attività commerciali, industriali e professionali. Dovremmo prevedere semmai un obbligo, senza alcuna diminuzione della tariffa, in

In ogni caso, l'approvazione di questo testo contro lo spreco alimentare è anche per noi un importante passo in avanti rispetto alla situazione attuale, anche se avremmo preferito una discussione in grado di accogliere il lavoro emendativo svolto da tutto l'arco parlamentare. Come Sinistra Italiana condividiamo l'importanza di colmare l'assenza ed ritardo che il nostro Paese aveva su questi temi e pertanto voteremo a favore del testo, anche se riteniamo che, in ogni caso, parliamo di un testo debole, proprio per l'assenza di obblighi specifici e direttamente verificabili e la non volontà di immaginare obiettivi più ambiziosi. Per noi gli ordini del giorno approvati oggi sono un impegno serio; verificheremo nel corso del tempo che il Governo

un provvedimento di grande importanza a nostro avviso, che reca disposizioni di rilievo indiscutibile, sia sul versante della lotta agli sprechi, sia sull'altro versante, altrettanto importante, che comporta il riconoscimento del lavoro straordinario che il terzo settore svolge, con varie attività di tipo assistenziale rivolte alle fasce più bisognose della nostra popolazione, per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari e farmaceutici con finalità di solidarietà sociale. Voglio anche dire, come Presidente della Commissione agricoltura, il lavoro in Commissione è stato molto positivo ed utile. Il dibattito in Assemblea oggi non ha reso pienamente lo spirito con cui da parte di tutte le forze politiche vi è stato un concorso a definire un *iter* rapido del provvedimento e a completare, attraverso ordini del giorno che oggi sono stati accolti, il disegno che il Parlamento, il Senato, vuole dare a questo problema. problema. È un provvedimento importante, che definisce un quadro normativo certo, che fornisce a sua volta una base legislativa solida ad attività di grande rilievo sociale, tuttavia svolte finora soltanto in maniera spontanea, senza un quadro normativo chiaro. Quando dico «spontanea» non intendo affatto qualcosa di negativo, al contrario: nella mia, nella nostra concezione c'è grandissima stima e apprezzamento per quei cittadini che, in maniera personale o associata, danno danno vita ad iniziative gratuite, con forte impegno delle loro capacità personali e del loro tempo per dare una mano alle persone - e sono tante in Italia - meno fortunate di loro. era importante dare un quadro normativo e questa legge finalmente lo dà. Definisce le modalità di cessione gratuità delle eccedenze alimentari, garantisce sia il cedente che il cessionario, fissa i requisiti per la conservazione delle eccedenze alimentari, fissa le garanzie sullo stato di alimenti, farmaci e altri prodotti nelle forme della distribuzione gratuita. Viene anche istituito un tavolo di coordinamento, con il coinvolgimento di un ampio numero di rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo. Viene rifinanziato il fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e viene creato un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze. Questo provvedimento affronta anche la materia della distribuzione di articoli di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale e per organizzare la raccolta di medicinali usati o scaduti per la donazione o o l'impiego. Assistono questi interventi norme di copertura e misure di favore a livello fiscale. L'approvazione, della quale sono certo, di questo provvedimento nello stesso testo stesso testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento consentirà l'immediata entrata in vigore del provvedimento e quindi consentirà di venire incontro tempestivamente alle pressanti istanze che vengono dal mondo associativo, dal terzo settore e, in ultima analisi, da un'ampia fascia della popolazione che beneficerà dei positivi effetti della normativa. Detto questo, qualche minuto ancora per approfondire due aspetti e fare un'operazione di verità rispetto a qualche luogo comune che ha circolato in queste settimane sulla stampa, anche su quella che si presume sia molto informata. Il primo aspetto di questo provvedimento riguarda la lotta agli sprechi. È importante che l'Italia, con questa legge, si doti, per prima tra i Paesi moderni, di un provvedimento organico su questo versante. Si è detto spesso in queste settimane ed ho letto da diverse parti che l'Italia sarebbe posizionata all'ultimo posto, come quadro normativo, rispetto alla lotta allo spreco alimentare. Non è così.

I dati del Politecnico di Milano, presentati all'Expo di Milano nell'ottobre 2015, dicono che ci sono 5 milioni di tonnellate annue di eccedenze alimentari recuperabili, di cui il 55 per cento lungo la filiera agroalimentare e il 45 per cento dei consumatori.

agendo sia sulla filiera agroalimentare per favorire la donazione di alimenti, sia sui consumatori con campagne di sensibilizzazione e di educazione che il provvedimento stesso prevede. In secondo luogo, come già accennavo nella prima parte del mio intervento, questa legge costituisce anche una grande possibilità di sostegno alle decine di migliaia di associazioni che si rendono disponibili a dare assistenza agli oltre 4 milioni di concittadini indigenti assoluti del nostro Paese. Come avverrà Colleghi, non è che prima di questa legge non ci fossero norme, ma nessuna era all'interno di una legge specifica contro lo spreco alimentare e questo causava difficoltà di utilizzo da parte dei donatori. Oggi invece, attraverso la chiarezza delle definizioni e anche dei termini di «operatori di settore alimentare», «soggetti cedenti» e «eccedenze alimentari», questa situazione di incertezza viene superata. Per i beni alimentari confiscati viene confermato che le autorità dispongono la cessione a soggetti *non profit*. Questa legge rende stabile l'incentivo ai donatori, già previsto dall'ultima legge di stabilità e che diversamente ogni anno doveva essere riconfermato. Queste ed altre note ulteriori, ad esempio il riconoscimento e l'incentivo del valore prioritario del recupero di cibi ed alimenti attraverso le donazioni per fini umanitari, fa sì che che io sia convinto che il Senato possa e debba votare con un ampio voto un provvedimento che ci colloca ai primi posti nel novero dei Paesi avanzati, per far fronte contemporaneamente a due battaglie: la lotta allo spreco e un'assistenza dignitosa e stabile ai nostri concittadini indigenti. *(Applausi in Italia più di quattro adulti su dieci sono in sovrappeso, un dato che riguarda tutte le fasce d'età, comprese quelle più tenere e che lievita, è proprio il caso di dirlo, ad una persona su due per chi si siede a tavola in Campania, Basilicata, Sicilia e Molise. Sono queste le recenti cifre diffuse dal sistema di sorveglianza dell'Istituto superiore di Sanità e qualcuno potrebbe chiedersi cosa c'entri tutto questo con gli sprechi alimentari. In realtà, sprechi, obesità e denutrizione sono gli assurdi anelli di una stessa catena, quella del paradosso alimentare. In un contesto globale dove la capacità produttiva oltrepassa il fabbisogno, se da una parte del mondo c'è un morto per denutrizione, dall'altra ne muore uno per sovralimentazione. Ed è assurdo pensare che mentre in quest'Assemblea - quella di una nazione evidentemente sovralimentata - si decide delle modalità di cessione delle eccedenze, in altri 33 Paesi fuori di qui, di cui 26 in Africa, vige una perenne insicurezza alimentare per via di siccità, alluvioni, conflitti civili. Una lista variegata che comprende Siria e Yemen, ma anche Niger, Camerun, Ciad e Repubblica Democratica del Congo, tanto per fare qualche esempio. Territori che ogni giorno accolgono rifugiati dai paesi limitrofi e che vivono la fase 3, fase 3, che i tecnici definiscono fase di crisi nutritiva e che è destinata a crescere secondo la FAO. Una raccapricciante geografia che investe anche i cambiamenti climatici, l'ambiente, la natura. Sì, perché è inconcepibile pensare che gli abusi perpetrati nell'agricoltura, nell'allevamento e nella pesca non abbiano conseguenze. Purtroppo le conseguenze esistono eccome e le paghiamo ogni giorno in catastrofi naturali. È importante prospettare una cultura alimentare alternativa, buona per la salute, amica dell'ecosistema. Partendo proprio dall'ambiente, esigiamo che nel contesto del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti si giunga non solo ad una semplice riduzione, bensì alla fine dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili. Considerati gli effetti negativi su salute e ambiente, dunque, chiediamo di favorire un'educazione alimentare che privilegi un ridotto impatto sull'*habitat* e sulle risorse naturali, con particolare attenzione alla diminuzione dei consumi di pasti di origine animale. necessaria chiarezza delle etichette. Per questo ribadiamo la necessità che siano esattamente indicati la data di scadenza e le condizioni di conservazione dei prodotti che costituiscono eccedenze alimentari. Non solo. I distributori automatici di prodotti alimentari devono recare all'esterno, in forma chiaramente leggibile, l'elenco dei prodotti e dei singoli ingredienti. Su tutti gli articoli alimentari e bevande potenzialmente dannosi per la salute, specie quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata, in modo chiaro e decifrabile, la dicitura «l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie». È fondamentale rendere cogente per gli operatori del settore la cessione gratuita delle eccedenze destinate agli indigenti, in ossequio ad idonee procedure di confezionamento, trasporto, distribuzione, deposito e utilizzo e nel rispetto della filiera corta e del benessere animale. I cessionari delle eccedenze, inoltre, devono osservare non solo le norme in materia di igiene e sicurezza alimentare, ma anche quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro. Chiediamo inoltre che con decreto del MEF, di concerto con il Ministro della salute, a decorrere dal 2016, i produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti debbano versare un contributo straordinario il cui ricavato andrà a beneficio dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito internet comunale per gli esercizi commerciali del settore alimentare che praticano l'autocompostaggio dei rifiuti organici, si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale, somministrano prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Esercizi, questi, che vanno premiati e incoraggiati con la destinazione di risorse aggiuntive. I Comuni, inoltre, proprio per favorire la filiera locale del riuso e per agevolare le donazioni, devono individuare idonei centri di raccolta per il deposito temporaneo dei beni alimentari che, in ogni caso, devono essere tracciati nel rispetto dei principi della rotazione, della trasparenza e dell'evidenza pubblica. Vanno poi previste delle sanzioni serie per chi dolosamente fa perire i prodotti alimentari eccedenti e ancora destinabili al consumo, con un'attenzione in più per il pane, accompagnatore indiscusso del companatico sulle nostre tavole. Gli enti che ricevono le cessioni gratuite devono avere precise caratteristiche e, cioè, devono avere statuti in cui sia riportata espressamente l'attività di beneficenza e devono essere iscritti in apposita sezione dell'elenco tenuto dal Ministero del lavoro o in un equivalente elenco regionale. Questa attività, infatti, se non censita e correttamente monitorata, rischia di generare situazioni non trasparenti che possono poi contrastare con la finalità della legge, vale a dire quella di ridurre per davvero lo spreco alimentare. È necessario porre un espresso divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private, nazionali o locali, nelle fasce orarie di programmazione rivolte ai minori e nelle ore destinate ai pasti, prodotti alimentari e bevande che contengono per noto un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, oltre che olio di palma, la cui assunzione eccessiva può essere molto dannosa per la salute. Occorrono, poi, percorsi educativi e formativi nelle scuole, al fine di ridurre e demotivare la somministrazione di cibi grassi. Per questo è opportuno promuovere la divulgazione di informazioni utili, linee guida, iniziative istituzionali e campagne informative sull'argomento e sullo spreco alimentare in genere. Il Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze deve avere dei destinatari virtuosi, ovvero chi fa del riutilizzo la propria eccellenza, specie per l'asporto di avanzi di cibo, chi promuove diete alimentari con prevalenza di prodotti di origine vegetale, anche in considerazione degli impatti poco ecologici connessi al consumo di carne. Il tutto deve avvenire attraverso procedimenti ad evidenza pubblica, anche nell'ambito della dichiarazione dei soggetti beneficiari di utilizzo dei beni ceduti, e con l'ausilio di un costante monitoraggio dei dati relativi allo spreco nella filiera agroalimentare. In tema di gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, è tempo che le pubbliche amministrazioni prevedano specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero e cessione gratuita delle eccedenze, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari più vicini al luogo di consumo e che dimostri di essere parte attiva nella riduzione a monte degli sprechi, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del *post* raccolto. Ribadiamo poi il coinvolgimento, nell'ambito della cessione gratuita di altri prodotti a fini di utilità sociale, anche degli enti pubblici, purché non perseguano finalità aventi scopo di lucro. Tutto questo può e deve accadere. Occorre ripensare questo tema in un'ottica multidisciplinare perché il cibo non è solo vita, è anche ambiente, salute e tutela dei diritti umani. Dichiaro, perciò, il voto favorevole del Movimento 5 Stelle con degli imprescindibili moniti. I ricercatori di Last Minute Market, lo scorso settembre, hanno ribadito che un terzo del cibo prodotto annualmente viene gettato nella spazzatura. Parliamo di oltre un miliardo di tonnellate di cibo, quattro volte la quantità necessaria per nutrire gli affamati del pianeta, stimati in 868 milioni di persone. Questo vuol dire che le produzioni normative non bastano; occorre sensibilizzare in maniera capillare l'opinione pubblica, le imprese e le istituzioni sul problema degli sprechi e sulla necessità e l'urgenza di ridurli, fino ad eliminarli. La grande distribuzione, le multinazionali, i colossi del cibo-spazzatura non possono continuare a girare la testa dall'altra parte. Concludo con una frase del padre della non violenza, vegetariano per scelta, guida spirituale per il suo Paese ed esempio per tantissime persone nel mondo. Quest'uomo, a ragione, affermava che l'arma più potente sulla terra è la forchetta. Mi riferisco a Gandhi. Ebbene, Gandhi sosteneva che la terra fornisce risorse sufficienti a soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l'avidità di ogni uomo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, normalmente la dichiarazione di voto si esprime alla fine dell'intervento, mentre io la esprimerò subito, dicendo che il Gruppo che rappresento voterà a favore

quanto per il fatto che non si sia voluto condividere un provvedimento che doveva essere supportato da tutti. Chi può dire di essere a favore dello spreco alimentare? Nessuno, ovviamente. Allora, se questi sono i principi che tutti condividiamo, perché non approvare

finalizzata, per qualche recondito motivo, a vantaggio di una categoria, bensì a vantaggio di quei consumatori che, giustamente, anche se meno abbienti, hanno il diritto di avere una figura qualificata, così che non si tratti di una prerogativa solo di chi paga il farmaco e, in quanto tale, fruisce già di questo servizio. Perché non prevederlo anche per le persone che veramente non hanno la possibilità di pagarsi i farmaci e che, attraverso questo provvedimento, un giorno ne potranno fruire? Reputo che non sia stato giusto, da parte del Governo, assumere un atteggiamento di chiusura. Non lo è stato, assolutamente, signor Vice Ministro. Non mi Non mi soffermerò nello sgranare dati di milioni di persone che muoiono di fame e, per contro, di milioni di persone che abusano del cibo al punto tale da morirne. È stato detto ampiamente, i principi sono stati enunciati, elencati e articolati in modo corretto. Ora vedremo come verranno poi applicati, nel momento in cui questo provvedimento dovrà avere anche operatività, perché altrimenti vuol dire che avremo fallito.

tante volte diventa quasi un sogno, perché poi, girandomi, non ho più visto il Ministro, dopo che ha fatto la sua dichiarazione, dicendo che bisogna perseguire questi risultati. Avrei voluto dire al Ministro, e dico a lei, signor Vice Ministro, che invece è molto presente e gliene do atto, a

perché non c'è più la convenienza a produrre. Non pensate che sia anche questo uno spreco alimentare? Non pensate che bisogna veramente mettere a punto una politica per far sì che questo o perlomeno che questa produzione e questi prodotti possano essere utilizzati a fin di bene? Anche acquisire

Aveva ragione il collega Candiani, quando sottolineava che siamo preda forse di una distrazione rispetto a ciò che accade fuori di qui. Aggiungo

nel dichiarare il voto favorevole e convinto del Partito Democratico, vorrei tornare su alcuni dei contenuti di questo disegno di legge, perché è un'iniziativa parlamentare promossa da 217 colleghi alla Camera, che ha unito dieci disegni di legge, e voglio ricordare quello della collega

convintamente, non senza discussione e dibattito, di non apportare modifiche al testo Camera, raccogliendo le numerose esortazioni che i soggetti auditi avevano rivolto in tal senso e anche raccogliendo in ordini del giorno diversi contenuti (penso al disegno di legge della collega Laura Puppato). È un lavoro che raccoglie anche quanto proposto dalla Commissione ambiente, all'unanimità, nel gennaio 2015, durante la discussione sul collegato ambiente, a proposito di semplificazione amministrativa per i soggetti donatori e di ampliamento della platea dei riceventi le donazioni. Non voglio dilungarmi sui dati e ne cito soltanto pochissimi, che riguardano il nostro Paese. Secondo l'osservatorio Last minute market, dell'Università di Bologna, lo spreco alimentare vale oltre 8 miliardi di euro, circa mezzo punto di prodotto interno lordo, pari a 800 euro a testa per ogni italiano. Parallelamente, come ha ricordato la relatrice, senatrice Bertuzzi, la povertà in Italia è cresciuta, tanto

provare a ridurre questa diseguaglianza e ad impostare un sistema economico circolare, che sprechi il meno possibile, soprattutto tra i beni primari come il cibo. Abbiamo bisogno di farlo subito, senza attendere ulteriori condizionamenti, soprattutto delle corporazioni, che anche in questa Assemblea abbiamo ascoltato essere eccessivamente presenti.

Ci sono tante persone, enti locali, università, associazioni di impresa, ONLUS, soggetti del terzo settore e della cooperazione (di consumatori), che hanno promosso in questi anni progetti importanti, sulla base della normativa del buon samaritano, certo, ma anche sulla base di mozioni, di indirizzi, di volontà politiche europee e nazionali. progetti nati già alla fine degli anni Novanta e agli inizi degli anni Duemila. Penso a quelli della mia Provincia, promossi dalla Coop di consumatori o dalla cooperazione sociale, chiamati con nomi particolari come «City cibo» o «Brutti ma buoni», ancora operativi, poi acquisiti a livello nazionale con nomi altrettanto significativi, come «Buon fine». Penso al ruolo svolto dalla Fondazione banco alimentare e dalla Caritas diocesana. Penso alla risoluzione

Penso allo *spin off* accademico della facoltà di agraria dell'università di Bologna promosso dal professor Segré, poi diventato laboratorio di riferimento nazionale ed europeo, con la nascita dell'Osservatorio nazionale sugli sprechi e con la definizione del primo Piano nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari. Penso all'associazione dei Comuni italiani «Spreco zero», fondata dal sindaco del Comune di Sasso Marconi e da Last minute market, per mettere in rete e implementare le buone pratiche e diffondere la cultura della lotta allo spreco. Accanto a tutto ciò, penso a ciò che ha significato l'Expo 2015 su questo tema e alle esperienze fatte in quei giorni nella mensa ambrosiana degli indigenti, per dimostrare, almeno in parte, che siamo quello che mangiamo. A proposito di Expo 2015 sono stati sottoscritti impegni solenni nella Carta di Milano, da tanti Paesi, tra cui anche il nostro, con il *premier* Renzi e il ministro Martina, a cui oggi diamo seguito in modo concreto e con un'iniziativa parlamentare. Proprio grazie ad Expo 2015 è risultato ancora più evidente a tanti come l'incremento dei consumi globali e dello spreco mettano sotto pressione gli ecosistemi in cui viviamo e come i problemi cruciali del pianeta, quali energia, ambiente, cambiamento climatico, povertà e cibo, non possano essere affrontati separatamente, ma quanto siano problemi sistemici, interconnessi e interdipendenti. Una circolarità che oggi l'Unione europea riconosce come strategica per lo sviluppo industriale e sostenibile del Continente ambiente, beni ambientali del Senato ha chiesto che includa anche una normativa unitaria contro lo spreco di cibo. Nell'attesa di quella definitiva scelta europea, il nostro Paese oggi decide di fare la sua parte, in modo originale, migliorando e innovando le disposizioni già vigenti, superando l'incertezza e gli ostacoli, dando un quadro organico per agire contro lo spreco alimentare e non solo, con una logica partecipativa e premiante. disegno di legge c'è stato anche quello di rendere effettivamente praticabile la destinazione a fini di solidarietà sociale dei prodotti non più vendibili e sottrarre tali prodotti allo spreco e alla distruzione, riducendo di conseguenza la produzione di rifiuti. Sì, rifiuti, perché il loro smaltimento costa mediamente 70 euro a tonnellata e la riduzione dello spreco di centinaia di migliaia di tonnellate farebbe risparmiare alla collettività costi assai rilevanti, riducendo contemporaneamente gli effetti dannosi per l'ambiente delle diverse tecniche di smaltimento degli stessi. Rifiuti che, per giunta, essendo confezionati, non potrebbero nemmeno essere conferiti alla raccolta del rifiuto organico, dove praticata. Quindi la riduzione della produzione dei rifiuti come scelta politica di sviluppo sostenibile, che anche in questo provvedimento viene inclusa in modo importante e fattivo. Stiamo parlando, certo, dei prodotti alimentari, ma anche dei farmaci e dei vestiti, così come degli altri generi di prima necessità. Tali finalità sono perseguite attraverso norme di semplificazione e incentivi delle vigenti disposizioni fiscali e dei tributi locali, mediante un'estensione degli enti beneficiari e delle categorie di prodotti essenziali ammessi alla donazione, con le misure legate alla riduzione del *packaging*, alle etichette e al *family bag* per la ristorazione, alla cessione dei prodotti agricoli in campo. Sul tema della donazione dei farmaci abbiamo ascoltato oggi un dibattito interessante, troppo condizionato però da interessi corporativi. Sul tema, credo che gli impegni che il Governo si è assunto con ordini del giorno specifici, che anche i colleghi hanno richiamato, siano importanti e indichino il percorso cui ricondurre il lavoro dei prossimi mesi, a partire dalla discussione che la Commissione igiene e sanità ha saputo svolgere sul disegno di legge presentato da diversi colleghi, come sostenuto dalle senatrici De Biasi e Bianconi. Per questo ci assumiamo oggi la nostra fetta di responsabilità, a testa alta e con orgoglio, e scegliamo un deciso cambio di passo per il nostro Paese, portando in approvazione una buona legge, che valorizza e sostiene chi già opera in questo campo. Sappiamo che da oggi in poi servirà qualcosa in più, sul piano della comunicazione e dell'educazione, come il disegno di legge prevede e sostiene, anche raccogliendo l'esortazione venuta dai promotori italiani della trentaseiesima Giornata mondiale della terra. Penso al disegno di legge sull'educazione al cibo, a prima firma della collega Pignedoli. Penso a una capillare campagna europea di educazione alimentare e ambientale in ambito europeo. Penso alla proposta per un nuovo anno europeo contro lo spreco alimentare, da individuare entro il 2025, per monitorare gli obiettivi di riduzione dello spreco. Anche così potremo misurare l'efficacia della via italiana della lotta allo spreco che oggi fa diventare il nostro Paese più inclusivo, più responsabile e più giusto verso il presente, ma soprattutto verso il futuro dei propri cittadini. Una scelta virtuosa e lungimirante, che i senatori del Partito Democratico voteranno, oggi più che mai, con convinzione e determinazione. *(Applausi dal Gruppo

La distinzione e il reciproco rispetto delle prerogative costituzionali di Governo e Parlamento in forma di leale cooperazione dovrebbero richiedere il rispetto della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi,

Mi chiedo cosa farete, se mai dovesse passare la riforma costituzionale, con quel nuovo articolo 70, assolutamente bizzarro e prolisso, che avete approvato. avete approvato. Ci troviamo di fronte alla violazione anche dell'articolo 97 della nostra Costituzione, ossia alla violazione palese

solo l'attribuzione dei giusti poteri ai giusti organi, secondo le giuste modalità. Il potere legislativo spetta al Parlamento e al Governo solo in casi straordinari di necessità e urgenza sulla base di criteri di omogeneità e riconoscibilità dei contenuti.

Sappiamo che la Corte costituzionale, a partire dalla fine degli anni Novanta - anche in questo caso, perdonate la vocazione maledettamente didattica di ricordare la giurisdizione della Corte costituzionale nega la reiterazione dei decreti-legge; considera la reiterazione di un provvedimento straordinario ed eccezionale in se stessa incostituzionale.

ha rivendicato il processo amministrativo telematico e la firma digitale come - cito *verbatim* un'espressione del nostro Presidente del Consiglio

perché continua a non applicarsi veramente, continua a rimanere in quella onirica categoria che piace tanto al nostro Presidente del Consiglio dei valorosi proclami. Ma mai come ora il problema esiste. Signora Presidente, colleghi, sappiamo tutti che la giustizia amministrativa ha un ruolo fondamentale nel nostro Paese, e non solo per la regolamentazione dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ma ma anche per gestire tutte le medie, grandi e anche piccole opere con criteri di celerità ed efficienza, che, se mal gestite, allontanano gli imprenditori, la crescita e il benessere economico. Tutti noi lo sappiamo perché abbiamo avuto esempi drammatici di imprese straniere che hanno tentato di radicare attività economiche nel nostro Paese e, dopo sequenze ininterrotte di ricorsi, tardivamente decisi o non decisi, hanno deciso loro di andarsene. Mai come in questo caso, quindi, è assolutamente indispensabile che l'applicazione di una norma esista in natura e non sia solo un onirico proclama, soprattutto perché tutto il resto d'Europa che ci circonda applica il processo telematico, informatizza il processo - e non solo amministrativo, ma anche civile e penale - e vi applica la firma digitale. Quel fiore all'occhiello i nostri *partner* europei se lo sono messo veramente. E aggiungo *en passant* - ma è un dato non irrilevante - che noi ci saremmo anche impegnati in Europa a fare lo stesso già molto tempo fa. Quindi anche in questo caso dobbiamo sottolineare un'inadempienza. alla quarta proroga di termini per l'applicazione del processo amministrativo telematico, che due anni fa il nostro Presidente del Consiglio ha dato per fatto, è una gravosa conseguenza politica, è una scelta profonda, una scelta di inefficienza. Noi tutti sappiamo - non ho bisogno di raccontarvelo, voi me lo insegnate - che una giustizia tardiva, sia essa civile, penale o amministrativa, è una giustizia negata e quindi una non giustizia, inutile per tutti; addirittura il Governo lo ha detto. Potrei citare *verbatim* - l'ho fatto in Commissione - le parole del Governo nella relazione annuale sullo stato della giustizia, in cui dichiara e si afferma che la non applicazione di criteri di informatizzazione che velocizzano il processo rappresenta una grande delusione per i cittadini e un allontanamento e un disamore della loro fiducia nella giustizia. Quindi, se il Governo lo sa, perché non lo fa? E questa è solo una parte. La seconda parte - devo dire, colleghi, assai più insidiosa - riguarda la scelta di inserire in Commissione alla Camera, in maniera proditoria, un po' intempestiva e truffaldina, un provvedimento in realtà importantissimo, che riguarda l'arricchimento delle piante organiche del Ministero della giustizia. Inserire nuove assunzioni al servizio dell'amministrazione della giustizia per ruoli non dirigenziali è una cosa buona e giusta. Però, prima di tutto lo si dovrebbe fare non scippando al Parlamento la possibilità di discuterne; secondariamente, se lo si fa e si sbaglia, inserendolo come articolo di un decreto-legge in un ramo del Parlamento alla fine del dibattito, lo si deve fare quantomeno con criterio, ossia spiegando chi ha chi ha la legittima aspettativa di ricoprire quanti e quali posti, sulla base di quali criteri oggettivi, secondo quale ripartizione percentuale, magari magari identificando i soggetti che hanno un'aspettativa ad essere assunti. In realtà questo decreto-legge, in maniera molto confusionaria e devo dire di un'opacità non perfettamente in buona fede (questa è l'impressione che ne abbiamo tratto in Commissione e ne abbiamo lungamente discusso), identifica un certo numero di posti potenzialmente liberi, che devono essere coperti per scorrimento, il che significa quell'enorme graduatoria nazionale, quell'immenso e purtroppo montante serbatoio della graduatoria nazionale degli idonei, che noi tutti conosciamo, oppure per concorso. Ma allora, colleghi, il Governo, in maniera assolutamente solitaria e senza averne discusso con il Parlamento, inserisce un provvedimento che meriterebbe un disegno di legge a sé stante, perché stiamo parlando di radicare posti di lavoro al Ministero della giustizia. E lo fa senza dedicarvi un provvedimento, senza interfacciarsi con il Parlamento, senza ascoltare quello che il Parlamento ha a dire e senza dirci come le quattro categorie identificabili, ossia gli idonei della graduatoria nazionale, soggetti menzionati in questo provvedimento, ma non collocati potenzialmente in queste assunzioni, i soggetti che rimarranno dall'eliminazione delle Province, ancora non avvenuta (abbiamo finanziato proprio ieri le Province), i soggetti potenzialmente assumibili *ex novo* i famosi soggetti tirocinanti, che tutti noi sicuramente ricordiamo, perché sono persone che hanno prestato dal 2011, secondo la legge n. 98 del 2011, un'attività e un servizio meritevole - lo ha riconosciuto anche il Sottosegretario - all'amministrazione della giustizia presso i tribunali e che hanno, loro sì, maturato una legittima aspettativa, ecco, noi non sappiamo quanti di questi soggetti, come e sulla base di quali criteri oggettivi potranno accedere ai concorsi. Anzi, noi non sappiamo nemmeno se questi concorsi si celebreranno, perché, se questi posti saranno ricoperti per scorrimento (e sicuramente di soggetti idonei nell'enorme graduatoria nazionale che ne sono e tanti), non sapremo nemmeno se esisteranno assunzioni innovative al di fuori e al di là della graduatoria. Tutto questo colleghi, consentitemelo, non è serio. Oltre ad avere difficoltà di copertura, come abbiamo chiesto e abbiamo evidenziato in Commissione, perché esisterebbe anche un articolo un articolo non irrilevante, l'articolo 81, che prevede che nuove disposizioni siano coperte da apposita posta di bilancio dello Stato. Ci è stato detto che esiste un fondo del Ministero della giustizia che potrà coprire queste assunzioni indeterminato - per gli anni 2016 e 2017. Vedremo, non ne siamo molto convinti. E poi, che cosa succederà? basta procedere per strappi. Lo dico molto serenamente ma con grande preoccupazione: è la seconda volta che diciamo sostanzialmente le stesse cose e non perché abbiamo un approccio arteriosclerotico all'attività parlamentare, ma perché purtroppo ci confrontiamo con gli stessi problemi e dobbiamo riscontrare sempre gli stessi errori, le stesse inefficienze e la stessa inefficacia dell'attività di questo Governo. Quindi, per questo motivo, noi speriamo che questo provvedimento si fermi qui.

il più è stato detto. È stato richiamato l'articolo 77, l'articolo 70, ma credo che la costituzionalità debba rispondere ad un requisito, quello della ragionevolezza e una cosa del genere non può essere considerata ragionevole. Stiamo parlando della quarta proroga di un provvedimento che è stato differito nella sua applicazione per quattro volte, un provvedimento che nasce siamo nel 2016 e lo proroghiamo di sei mesi, un emendamento della Camera richiede altri tre mesi di proroga, per cosa? Per la realizzazione del processo amministrativo telematico. A me sembra evidente che il processo amministrativo e gli altri parenti del processo amministrativo siano esclusivamente il solito annuncio, che qualcuno ha voluto fare dicendo: d'ora in poi tutto viaggerà in formato elettronico. E questa è una presa in giro. Lo dico testimoniando una mia esperienza. Ho presentato un quesito referendario per l'abrogazione della legge Fornero: avendo raccolto 600.000 firme per potere sostenere

Leggo un giorno, sulla *Gazzetta Ufficiale*, che è stata convocata la seduta dove si dovrà decidere se è ammissibile o meno il *referendum*. Non avendo mai ricevuto alcuna notifica da parte della Corte costituzionale, mi reco presso la Corte per chiedere motivo della mancata notifica e gli uffici, scusandosi, fanno una ricerca e la raccomandata giaceva,

allora di cosa stiamo parlando: se la Corte costituzionale non è dotata della posta elettronica certificata, noi pretendiamo che il più lontano e minuscolo

Ci siamo resi conto, dopo che abbiamo abolito l'utilizzo del *fax*, che molti uffici non ne erano dotati. E noi adesso, ancora una volta, stiamo chiedendo una proroga? A me sembra che ci troviamo di fronte ad una presa in giro.

Si sfrutta quindi il passaggio alla Camera, e mi chiedo come la presidente Boldrini possa aver dichiarato ammissibile quell'emendamento e anche come il presidente del Senato

L'emendamento introdotto alla Camera dei deputati consente l'assunzione di mille unità di personale per i processi civili, penali e amministrativi; ma noi stiamo parlando di processo amministrativo; quindi, le sedi penale e civile non c'entravano assolutamente niente con quello di cui stiamo parlando.

fosse stato costituzionale, avrei votato una questione pregiudiziale rispetto alla costituzionalità perché si aggira il principio che si entra in un ruolo pubblico attraverso un concorso. Mille sono infatti i posti che andiamo ad assegnare - sembrerebbe una cosa bella - attraverso lo scorrimento di graduatorie di concorsi già realizzati - ricordo che c'è il ruolo unico e, quindi, non riguarda solo il settore giustizia, ma tutta la pubblica amministrazione e, quindi, prima si mettono a posto con lo scivolamento le attuali graduatorie e dopo si fa un concorso e si dice che si possono eventualmente considerare i titoli di coloro che hanno fatto il tirocinio presso le procure e i tribunali.

Decine di migliaia sono quelli che hanno fatto il concorso su Roma. Ma allora, dov'è il concorso? Sappiamo già che il concorso non si farà mai, che nessun posto verrà riservato a quelli che per 400 euro al mese fanno il tirocinio da dieci o vent'anni. Sappiamo che i nomi di quelli che verranno assunti

Chiedo e continuerò a chiedere che venga indicata la provenienza perché mi risulterebbe strano vedere collocato a fare il cancelliere in un tribunale

Grazie

è entrata a gamba tesa sulla vicenda delle assunzioni, che non c'entrava proprio nulla con questo decreto. Pertanto, voteremo a favore della questione pregiudiziale.

Presidente, non le nascondo che anche io sono stato colto di sorpresa, perché era previsto (perlomeno, così mi avevano informato) che la discussione generale si sarebbe aperta domani.

domani, se non direttamente stasera al termine della discussione generale. Siamo alle solite: il Governo

maggioranza e opposizione porta di fatto al varo di provvedimenti, mi lasci dire, perlomeno incompleti e certamente non esaustivi.

era nato con l'intento di snellire i tempi e le procedure del processo amministrativo telematico, e invece si è trasformato in una sorta di ufficio di collocamento che il Governo utilizza per incrementare

per questo e per altri motivi che sicuramente verranno meglio espressi nella dichiarazione

delle attività del Senato. Ciò perché bisogna produrre dei provvedimenti che siano il più possibile in linea con una crescita economica che il Paese si aspetta, dando di conseguenza alle imprese anche la possibilità di avere una più giusta, più equa e più rapida giustizia, anche se amministrativa. Così non è, perché i tempi medi

per gli investitori, che di certo non possono ritenere il nostro un Paese in cui agevolmente si riescono a fare

non è la scelta più giusta che il Governo avrebbe potuto fare, ma in realtà è quella che noi siamo soliti vedere, ossia un Esecutivo che preferisce twittare l'ennesima notizia, cioè dire «mille posti di lavoro in più»,

Presidente, vorrei farle notare che, in assenza del Governo, mi sembra che non ci sia più la possibilità di continuare questa discussione. Penso che la discussione generale su questo provvedimento, con tutta la nostra buona volontà, non possa proseguire in queste condizioni.

Signora Presidente, non sarei intervenuto se non reputassi il fatto grave. A volte può capitare anche ad uno dei maggiori e più prestigiosi quotidiani nazionali dei maggiori e più prestigiosi quotidiani nazionali la pubblicazione di un articolo che, pur trattando questioni particolarmente Grazie Grazie sui casi degli ultimi anni di violenze perpetrate in diverse forme contro bambini, in particolare in asili e scuole di diverse città italiane, tra l'altro compiute dai soggetti

potrebbero anche essere insite in non meglio precisate usanze e radici culturali. Parlando di quei fatti terribili, il dottor Zunino scrive Zunino scrive infatti: «Non sale dalla profonda Barbagia il racconto del maltrattamento dei piccoli alunni. Tocca Roma, Grosseto, Pisa, Bolzano». Non credo che si possa neppure evocare il rispetto della libertà di stampa, perché qui certamente nulla c'entra la libertà di espressione di un giornalista. Scritto così, quell'articolo è una perfetta fotografia razzista, fatta da un intellettuale - come è un giornalista - che propone nel nostro Paese discriminazioni tra gente che, per cultura, può fare cose orribili e gente che, per cultura, non dovrebbe farle. È un'offesa non solo agli abitanti della Barbagia, ma a tutta la Sardegna e ad ogni sardo. In Sardegna, ovviamente, da questa mattina l'articolo ha già generato molte polemiche e il direttore di Repubblica, il dottor Calabresi,

bisogna prendere atto delle scuse di quest'ultimo e pensare ad un tragico scivolone, come lui stesso lo ha definito. Mi permetto però di dare qualche brevissima informazione al dottor Zunino. La Barbagia è una vasta Regione montuosa della Sardegna centrale, che copre un'area di quasi mille chilometri, con oltre centomila abitanti. I barbaricini discendono dalle popolazioni prenuragiche e nuragiche, che sono tra le prime civiltà del Mediterraneo. Né i cartaginesi prima, né i romani dopo riuscirono a piegare la fierezza di quelle popolazioni. I romani li chiamarono «barbari» e da qui il nome di «Barbagia», che deriva dal latino *Barbaria*, appunto, per contrapporlo alla *Romania* e cioè il il resto del territorio che invece era sottomesso a Roma. Già da allora non si trattava di popolazioni selvagge o barbare, ma di popolazioni che fieramente non si fecero mai piegare completamente da Roma. Escludo che ci sia mai stata una cultura di violenza sui bambini. Non conosco personalmente il dottor Zunino,

sulla Barbagia, sulla sua storia, sulle sue tradizioni e sulla civiltà dei suoi abitanti. Certamente in futuro, almeno mi auguro, smetterà ed eviterà di scrivere sciocchezze come quelle che ha scritto questa mattina. *(M5S)*. Signora Presidente, noi siamo qui in Parlamento come portavoce dei cittadini, perché sappiamo benissimo che i cittadini normalmente subiscono, ma non hanno assolutamente la possibilità di avere voce. Pertanto, in questo momento mi faccio carico di questa anomalia.

c'è stata proprio una coercizione forzata di questo canone RAI, con il pagamento del canone attraverso la bolletta elettrica.

Presidente, io mi faccio carico di questo. Sarebbe opportuno che il Governo varasse immediatamente un provvedimento che consenta a queste persone che non hanno potuto pagare il canone a luglio di poterlo dilazionare

al Parlamento, ha anticipato, replicando poi questa posizione anche a Potenza, che l'ambientalismo lucano è oggetto di monitoraggio continuo da parte di Grazie un atteggiamento intenzionalmente finalizzato a screditare e criminalizzare. Invece in Basilicata, sempre per voce non più di Alfano, rappresentante delle istituzioni

indicato nella Basilicata una regione in cui le cosche della 'ndrangheta calabrese avevano effettuato, e stanno effettuando, massicci investimenti, probabilmente in operazioni che confliggono con il diritto ambientale e quindi con le battaglie poste in essere appunto dalle associazioni cui ho dato voce. A fronte di questo quadro, cosa fa il titolare del Viminale? Piuttosto che monitorare con maggiore attenzione come è stato dimostrato, delinque, chi oltraggia l'ambiente oltre che la salute delle persone, monitora appunto cittadini che, riunendosi in associazioni, cercano di

Al contrario, io auspico che associazioni di cittadini sempre più convinti della necessità di battersi contro uno Stato che rivela molto spesso una vocazione autoritaria e non democratica siano sempre più forti